Il Senato*,* in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», premesso che:

e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Le macroaree di intervento del Governo sono quattro e, in estrema sintesi, il contenuto è il seguente. La prima area è la funzione del turismo, che è trasferita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il primo si chiamerà Ministero dei beni e delle attività culturali, il secondo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo. La seconda area riguarda la funzione in materia di emergenza ambientale e di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche; è trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La terza area riguarda le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità ed è attuata e organizzata dal Ministero per la famiglia e le disabilità e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella quarta area è previsto, infine, il riordino di altre funzioni in materia di edilizia scolastica ed edilizia di emergenza. Entrando nel dettaglio, il decreto-legge si compone di cinque articoli. Il primo trasferisce, sin dalla entrata in vigore del decreto-legge, la competenza in materia di turismo dal MIBACT al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa la gestione residui, della direzione generale turismo. Il comma 2 del medesimo articolo, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, prevede la soppressione della Direzione generale del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e istituisce il Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole. Il comma 3 adegua e coordina il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alle novelle previste dai commi precedenti. I commi 4 e 5 prevedono l'adeguamento automatico, ovunque ricorrano, delle rispettive denominazioni dei Ministeri coinvolti. Il comma 6 prevede la modifica della denominazione e delle funzioni della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, in Scuola dei beni e delle attività culturali, lasciando al MIBAC le relative attribuzioni e le risorse necessarie al suo funzionamento, indicando il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per modificare lo statuto della Scuola. Il comma 7 attiene al personale. Entro quarantacinque giorni dalla conversione in legge del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si deve procedere ai trasferimento del personale e delle risorse.

e, comunque, dei progetti o convenzioni da essa stipulati. Il comma 8 prevede che il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale presso il MIBAC resti inalterato. Pertanto, a seguito delle modifiche, dispone l'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, il cui costo è compensato dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale non generale finanziariamente equivalente. Dispone poi che, con decreto del Presidente della Repubblica, il Governo adegui le dotazioni organiche del MIBAC e del Ministero delle politiche agricole e forestali. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede, al comma 1, il trasferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale, volti a garantire la sicurezza alimentare in Campania e il monitoraggio, anche di tipo sanitario, in Campania e nei comuni di Taranto e Statte. Il comma 2 dispone una serie di modifiche normative, in relazione a quanto stabilito al comma 1, prevedendo che la presidenza del Comitato interministeriale e della Commissione per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale in Campania siano di appannaggio del Ministero dell'ambiente.

disponendo conseguentemente alcune modificazioni testuali tra cui la soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio ItaliaSicura. Il comma 4 aggiunge una funzione a quelle del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse e coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino della sicurezza dei siti inquinati. Il comma 5 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie necessarie. comma 6 predispone le necessarie coperture per l'anno 2018 mediante la riassegnazione delle risorse allocate dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'ambiente e per il triennio 2019-2021 rinvia alla legge di bilancio. L'articolo 3 prevede il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità. Attribuisce alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministero per la famiglia e la disabilità, una serie competenze in materia di: politiche per la famiglia nelle sue componenti problematiche generazionali e relazionali; funzioni di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia; interventi per il sostegno della maternità e della paternità; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica; attività concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. In questo ambito, la Presidenza del Consiglio esercita: la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi previsti in materia. Sono inoltre attribuite, secondo le predette modalità, anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri e le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Sono altresì attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, in alternativa, al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore di persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità. Il comma 2, al fine di favorire le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, apporta modificazioni alla legge di stabilità del 2016 in materia di Carta della famiglia, prevedendo che l'eventuale adozione di nuovi criteri e modalità di rilascio della stessa sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, in alternativa, del Ministro per la famiglia e la disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Il comma 3 riconduce l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio. Il comma 7 dispone una riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 per garantire l'attribuzione di pari risorse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'articolo 4 va a novellare la normativa relativa all'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto Casa Italia e agli interventi di edilizia scolastica, e attribuisce e riordina altre competenze. Il comma 1 elimina la previsione che istituiva con legge un apposito Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 dispone che le risorse gestite dal soppresso Dipartimento e destinate ad interventi di ricostruzione nei Comuni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella zona Il comma 3 dispone modifiche alla legge di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019. In particolare, si trasferisce dalla Presidenza del Consiglio (Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la funzione di ricevere dagli enti locali la comunicazione degli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica.

la 1a Commissione ha esaminato per le parti di competenza il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. L'uso dello strumento del decreto-legge - e questo, signor Presidente, glielo vogliamo sottolineare in quanto lo riteniamo assolutamente importante - ha costretto la Commissione ad esaminare il testo con termini molto brevi, limitando enormemente la possibilità di sviluppare proprio in Commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. Tanto che - lo sottolineo più volte - l'opposizione non ha capito molte delle scelte che sono state fatte, perché non c'è stata la possibilità di discuterle. L'istruttoria legislativa in Commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata su un oggetto, come quello dell'organizzazione e delle attribuzioni dei Ministeri, che - lo ricordo per chi se lo fosse perso - sono esplicitamente assegnati alla legge dalla Carta costituzionale, quindi spettano ai parlamentari e alle Commissioni. Stupiscono le forze politiche dell'attuale maggioranza, che avevano promesso anche in quest'Aula al momento dell'insediamento, anche aderendo alla recente riforma del Regolamento del Senato, una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità, altrettanto importante, dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa. Ebbene, ci sembra invece di assistere ad un abuso, senza alcun pudore, della decretazione d'urgenza non utile, inadatta, in palese violazione del dettato costituzionale.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 L'attività della Commissione, ci dispiace dirlo Presidente, è diventata così molto frettolosa. Le audizioni si sono ridotte ad un'unica mattinata, molto sommaria, e l'Aula oggi è costretta ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti. che, anche rispetto agli emendamenti che andremo poi a discutere, sia stato fatto un approfondimento da parte di tutti i colleghi perché mancano quelle valutazioni rispetto alle proposte alternative che noi abbiamo continuamente fatto e con forza, a partire dalla pregiudiziale, che solo un serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono invece assicurare. In tale quadro, però, sono emerse rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge, quei presupposti - ricordiamo che il decreto-legge agisce quando ci sono delle necessità e delle urgenze - di necessità ed urgenza indispensabili per il suo legittimo utilizzo. Dove sono? Noi qui non li abbiamo proprio trovati e non è sufficiente, ci dispiace dirlo, la mera dichiarazione di necessità ed urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge se come, invece, in questo provvedimento in esame, il contenuto del decreto risulta assolutamente carente dei requisiti prescritti all'articolo 77 della Costituzione. Nel decreto-legge in esame, quindi, non vi è alcun riscontro oggettivo proprio di questa necessità ed urgenza, nelle disposizioni di cui ai primi tre articoli, dove viene infatti solo enunciata. Con riferimento all'articolo 1, il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, secondo quanto si legge chiaramente nella relazione tecnico-normativa, servirebbe favorire un rapido avvio di una politica integrata di valorizzazione del *made in Italy*. È una motivazione del tutto inconsistente che mostra, al contrario, come il trasferimento avrebbe potuto agevolmente essere contenuto in un normalissimo disegno di legge ordinario. Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, la necessità ed urgenza che dovrebbero giustificare l'inserimento delle norme nel decreto, non è in alcun modo motivata e, per quanto riguarda Il riordino delle attribuzioni dei Ministeri non è certo un evento straordinario, tanto che la definizione delle attribuzioni dei Ministeri - l'ho già detto prima e qui lo ribadisco

Governo ha una chiara e precisa volontà di espropriare il Parlamento delle sue competenze legislative. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, la ragione sottesa all'articolo 1 - lo dico ma, se ci fosse stato più tempo di dibattere, magari lo avremmo anche capito - che prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo in materia di turismo risulta assolutamente incomprensibile, considerato che, in questo modo, viene meno il legame, fondamentale per il nostro Paese, tra turismo e cultura. Risulta Risulta altrettanto poco credibile, non ci stancheremo mai di dirlo, definire il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - così come ho letto prima ed è descritto all'interno della relazione tecnica - Ministero del *made in Italy* Italy* per il semplice motivo che se l'intenzione del Governo fosse stata davvero quella di inserire il turismo tra le materie strategiche per lo sviluppo economico del Paese, il Ministero di riferimento sarebbe dovuto essere, naturalmente, dello sviluppo economico, come conferma, oltretutto, l'allocazione della materia del turismo presso le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica cui fa riferimento lo sviluppo economico. E, non a caso, signor Presidente, era una delle nostre proposte presentate come alternativa a quanto previsto dal decreto-legge. Infatti, prevedevamo il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di turismo, proprio perché almeno avremmo capito le motivazioni e saremmo stati assolutamente aderenti addirittura alla relazione illustrativa e tecnica; cosa cosa che oggi non è. Infine, il motivo per trasferire la competenza del turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non può neppure risiedere nelle personali competenze del Ministro che - lo ricordiamo - è pur sempre Ministro *pro tempore*. Sarebbe del tutto illegittimo decidere le attribuzioni e, conseguentemente, l'organizzazione di un Ministero e l'allocazione delle risorse dello stesso, sulla base delle presunte competenze di un Ministro nel quadro di una logica meramente spartitoria, a nostro avviso, dei poteri all'interno di una composita, ma alquanto equilibrata, maggioranza parlamentare. Nel senso che sulle spartizioni non vi batte nessuno. Si auspica quindi un'ulteriore riflessione sulla questione in esame, al fine di evitare una riorganizzazione che risponde ad esigenze politiche - e questa è la vera preoccupazione - più che all'obiettivo di garantire un ordinato ed efficiente assetto istituzionale. L'articolo 2 mette mano alle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo attribuiscono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia

la struttura di missione sull'edilizia scolastica. Soppressioni che non riusciamo a comprendere, considerato che si trattava di strutture efficienti, capaci di effettuare raccordi e coordinamenti tra enti e amministrazioni locali.

Per quanto riguarda l'utilizzo di questo strumento, che dovrebbe operare nel perimetro dell'urgenza, molti colleghi hanno già avuto modo di esprimere le giuste obiezioni che, condividendole, non riproporrò nel mio intervento. Sorvolerò invece per motivi di tempo sul fatto che se è vero che questo provvedimento ridisegna le competenze sui vari settori e dipartimenti, è altrettanto vero che il testo in esame non ci mette un centesimo di euro. Questo ci porta a dover credere, ad esempio, che le competenze del turismo in capo all'agricoltura attiveranno un maggior giro di affari per il settore, convinzione però a cui dobbiamo abbandonarci sulla fiducia, non essendo specificato come, quando e perché. In particolare, trasferire a un apposito Dipartimento del Ministero delle politiche agricole le funzioni in materia di turismo, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie e le necessarie modifiche normative conseguenti, riguardanti gli enti vigilati, sembra muoversi nella direzione di svilirne l'importanza. Per questo, oltre alle eccezioni che seguiranno, merita di essere affrontata anche la questione legata ai segnali che vogliamo mandare all'interno e all'esterno delle nostre istituzioni e del Paese. Quello che ci si dovrebbe aspettare da un Governo del cambiamento è come minimo il superamento, in maniera articolata, di ogni ostacolo o resistenza, come quello della burocrazia della burocrazia. Invece, purtroppo, ci troviamo di fronte a un provvedimento che porta in dote i soliti problemi relativi ai dipendenti ministeriali da trasferire di Ministero in Ministero, senza che si parli mai di produttività o almeno di progettualità. Ancora: le competenze che riguardano il turismo, ora accorpate al Dicastero dell'agricoltura, inducono a fare alcune riflessioni. Brevemente, ricordo ai colleghi che il Ministero del turismo e dello spettacolo fu istituito nel 1959, poi abrogato nel 1993 e poi di nuovo ricostituito dal Governo Berlusconi nel 2009, l'unico Governo con la lungimiranza di capire che un Paese come l'Italia, sul cui PIL il turismo incide per oltre il 12 per cento, ha bisogno di un Ministero del turismo. E guardate, non lo dico per essere polemico, ma, se ci si assume l'onere e l'onore di rappresentare i cittadini e ancor più di governare questo Paese, c'è bisogno di coraggio, non della paura, della fragilità e dell'incertezza di questo Governo, che dichiara di voler trasferire delle competenze da un Ministero a un altro, per poi un giorno forse dare al turismo la dignità di Ministero a sé, che invece meriterebbe. Ciò che manca, ora più che mai, è la perspicacia di guardare al futuro e ai provvedimenti da attuare, in un ottica *a priori* e non *a posteriori*. Quello che ci si aspetterebbe dal Governo del cambiamento e della partecipazione è che ci si attenesse a quanto sottoscritto nel contratto di Governo, che riporta, al punto 26, gli indirizzi per il turismo. Cito testualmente: «Un Paese come l'Italia non può non avere un Ministero del turismo, che non può essere solo una direzione di un altro Ministero, ma ha bisogno di centralità, di *governance* e di competenza, con una *vision* e una *mission* coerenti ai grandi obiettivi di crescita che il nostro Paese può raggiungere». Questo è scritto nel contratto di Governo. Allora mi chiedo e chiedo al Governo: dobbiamo avvalorare la tesi che questo passaggio al Ministero delle politiche agricole sia per dare un senso alle competenze del Ministro? Se così fosse, allora, soprassedendo bonariamente sulle ritualità della scelta, che si istituisca il Ministero del turismo, con a capo il ministro Centinaio. La posizione di questa opposizione, la posizione di Forza Italia è chiara e decisa, e sono i dati a indicarcela. Il turismo - lo ricordavo prima - vale oltre il 12 per cento del prodotto interno lordo e ha un peso più che rilevante sull'economia del Paese, con circa due milioni e mezzo di cittadine e cittadini che lavorano in questo settore, animato da oltre 650.000 imprese. Il prodotto interno lordo dell'agricoltura, di contro, è sceso - ahimè - a 28 miliardi nel 2017 ed è stato l'unico settore che ha registrato un calo pari al 4,4 per cento e un -1,2 per cento sull'occupazione. A questo punto è naturale chiedersi se, addirittura, un accorpamento del turismo nel Dicastero dell'agricoltura non possa comportare un rallentamento di un settore, come quello del turismo, che al contrario ha registrato un'ottima crescita. Il turismo non è solo agriturismo, come l'agricoltura non è e non potrà mai essere solo agriturismo. Farli incontrare è una buona idea, ma confonderli significherebbe non avere idee. Sappiamo che l'Italia vanta, in tutte le nostre Regioni, un patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, frutto delle numerose civiltà fiorite nei millenni sul nostro territorio e nella lunga e perdurante interazione tra uomo e natura. Sappiamo che la cultura dell'accoglienza italiana è indiscutibile e non parlo solo di albergatori e ristoratori, ma di tutti gli esercenti che vivono quotidianamente nei nostri borghi, nelle nostre metropoli e nelle nostre città. Credo che ci sia bisogno di una svolta, dunque, che rafforzi l'Italia come museo diffuso; che abbia la forza di proporre nuove destinazioni ai turisti stranieri e che rilanci la *leadership* nel nostro Paese sul mercato mondiale, come epicentro del turismo sostenibile e di qualità, in grado di essere strumento di benessere economico e sociale per tutti. Bisogna tenere presente poi che la composizione della spesa dei viaggiatori è cambiata e vede, sì, in rilevante aumento l'importo per l'alloggio, ma anche quello dei servizi connessi. Pertanto, si dovrebbe puntare su nuovi accordi commerciali con l'estero e aiutare, con veri piani strutturali, le imprese che offrono servizi aggiuntivi per i nostri turisti, che invece, ad oggi, sostengono da sole questi investimenti che fanno bene al Paese. Il modello di sviluppo che andrebbe immaginato per il turismo dovrebbe proporsi come puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse, secondo un modulo di interdipendenza orizzontale, recuperando, anzi rivalutando, in un ambito territoriale a diversi livelli non omogeneo come il nostro, il coinvolgimento attivo di operatori e utenti. Ovvero, la sfida che si trova ad affrontare oggi il settore del turismo è ambiziosa: governare un sistema complesso di offerta in un mercato sempre più dinamico e in rapida e costante evoluzione, cercando di affermare la *leadership* dell'Italia come il Paese per eccellenza che i viaggiatori amanti di arte, cultura, moda, ambiente ed enogastronomia dovrebbero visitare. E come può essere vinta se non con un Ministero che si occupi solo di questo? Lo abbiamo già significato al ministro Centinaio: il comparto agricolo, fondamentale per il nostro Paese, soffre già di annose questioni e problematiche strutturali, a cui andrebbe dedicata la sua totale attenzione. Non credo, quindi, che possa trovare il tempo le risorse, per occuparsi di una delega che resta troppo distante da questo settore. A meno che, s'intende, non pensi che per poter promuovere il turismo italiano bastino i suoi cinguettii nell'etere. Basta con i tentennamenti. Se anche il Governo crede di voler arrivare all'ovvia necessità di istituire un Ministero del turismo, che lo faccia adesso e non ci costringa a questo avvilente spettacolo della politica del cambiamento, che vive in differita fra un contratto, un annuncio e il suo contrario. apre una nuova finestra") *(PD)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, giudico molto importante questo provvedimento, a differenza di quanto

il quale, con voce commossa, spiegava che in quel momento egli stesse scrivendo la storia. Ora noi abbiamo perso un po' il ritmo perché la rapidità e l'intensità con cui il Governo sta scrivendo la storia sono sinceramente degne di nota, per noi *demodè*, la storia la scrivono i Churchill e i Mandela, dobbiamo abituarci a pensare che, per altri, la scrivono i Costa e Di Maio. *(Applausi dal Gruppo PD)*. L'elemento chiave di questo provvedimento, secondo il ministro Costa, stava nell'attenzione ai temi ambientali. Lascio qualsiasi argomentazione sul Ministero del turismo e su quello della disabilità e mi limito a considerare e a lasciare agli atti di questo Parlamento, non ancora obsoleto, la considerazione su ciò che è stato fatto in questi quattro anni. Con questo Governo e con questo decreto-legge si mette la parola fine alle unità di missione denominate ItaliaSicura. Questo decreto-legge non mette un centesimo in più di denari sull'edilizia scolastica o sul rischio idrogeologico; se questo avvenisse, noi saremmo i primi a fare l'applauso alla maggioranza. ci sarà un aumento di denari nei settori dell'edilizia scolastica e della lotta al rischio idrogeologico, noi staremo dalla vostra parte. Ma non avete fatto questo, signori del Governo, cui mi rivolgo per il tramite del signor Presidente del Senato: voi avete cancellato delle strutture, nate quattro anni fa, come primo gesto del nostro Governo, strutture che hanno in pancia cantieri per 9 miliardi in un caso e per 7 miliardi in un altro, strutture rigorosamente *bipartisan.* Chiedetelo al Presidente della Regione Liguria se l'unità di missione ItaliaSicura è stata utile per il Bisagno. E vi garantisco che il Presidente della Regione Liguria non è un pericoloso compagno o un sovversivo comunista. Chiedetelo agli amministratori locali della Lega, come di tutti gli altri schieramenti,

Allora, il ministro Costa ha fatto la storia cancellando queste unità di missione. Vorrei semplicemente dire che non condividiamo questa scelta. Lo vorrei dire senza alcun tono polemico, ringraziando chi ha lavorato in questo settore, le donne e gli uomini, gli ingegneri, geometri, architetti e muratori che hanno lavorato in questo settore in questi anni, e dicendo che si è persa un'occasione. Chi, dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, ma anche delle opposizioni, era in quest'Aula nella scorsa legislatura - io ci sono stato soltanto dalla parte del Governo e non per tutta la legislatura - ricorderà, lei lo sa, signor Presidente, che non è stata una legislatura particolarmente distesa nei toni tra le opposizioni e la maggioranza di allora. C'è stato soltanto un momento, perlomeno nei tre anni in cui ho avuto una qualche responsabilità in cui, per merito di tutti, il clima è stato tranquillo e condiviso. Mi correggeranno i colleghi che erano senatori anche nella scorsa legislatura: per me è stato quando ha parlato in quest'Aula Renzo Piano, che ha raccontato il progetto Casa Italia e ha ricordato a tutte e a tutti noi che quel progetto aveva bisogno di un orizzonte temporale ultradecennale per dispiegare i suoi affetti. Tutte le forze politiche hanno detto in quel dibattito: sì, manterremo Casa Italia chiunque vinca le prossime elezioni. In questo decreto-legge, in cui si fa la storia, Casa Italia viene cancellata e io penso che sia un'occasione persa, innanzitutto per i nostri figli. Amici della Lega, permettetemi di dirvi con una battuta che avete utilizzato la ruspa nella direzione sbagliata! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avevate immaginato, proclamato e vinto le elezioni dicendo che avreste demolito la legge Fornero, ma avete demolito le unità di missione sulla scuola e sul rischio idrogeologico. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dovevate fare il reddito di cittadinanza e fate il decreto disoccupazione; dovevate bloccare le tasse, ma state bloccando l'ILVA. Penso che questo dibattito non faccia la storia. Noi, al massimo, le storie le possiamo fare su Instagram, non abbiamo la forza del ministro Costa, ma può essere importante per mettere dei punti fermi. Oggi il Presidente del Consiglio è a Washington e alla Casa Bianca, davanti al Presidente degli Stati Uniti d'America, dirà sì al TAP, forse domani un qualche ex parlamentare da una piazza del Guatemala dirà di no al TAP davanti a YouTube. Oggi il ministro Salvini darà la solidarietà ai carabinieri e ai poliziotti aggrediti nei cantieri TAV e noi saremo col ministro Salvini quando darà la solidarietà ai carabinieri e ai poliziotti aggrediti nei cantieri TAV. E vorremmo essere con il ministro Salvini quando darà la solidarietà a quei cittadini italiani dal colore della pelle diverso che vengono aggrediti in queste ore con qualcuno che dice che non c'è emergenza. Vorremmo dare la solidarietà al ministro Salvini quando si schiera da quella parte, ma anche sulla TAV ci sarà un altro Ministro che si concentrerà e dirà no, dobbiamo ancora decidere. Allora, signor Presidente del Senato, stiamo vivendo una fase strana, nella quale certe scelte incidono e incideranno sul futuro delle nostre storie e delle nostre vite. Penso che questa maggioranza abbia tutto il diritto di scegliere le persone che ritiene nei luoghi per i quali la legge prevede che si possano scegliere ad esempio, nelle unità di missione la maggioranza avrebbe avuto la possibilità di indicare nuove professionalità, non è la presidenza della RAI, dove per legge occorre avere una maggioranza più alta di quella che sostiene il Governo e se si indica alla presidenza della RAI uno che ha come caratteristiche personali quella di parlare male del Presidente della Repubblica, di essere contro l'Europa, di mettere in discussione i vaccini, poi non ci si può stupire che, a norma di legge, noi diciamo di fare senza di noi. Non ci si può stupire di questo. *(Applausi dal Gruppo PD).* In questo caso, però, sarebbe bastato scegliere un nome autorevole e il Governo avrebbe potuto indicare un nuovo responsabile per l'unità di missione. Non è accaduto, signor Presidente, signor Presidente, e oggi quella che è stata la nostra prima scelta, con il sottosegretario Delrio, fare due unità di missioni, una per la scuola e una per il rischio idrogeologico, diventa la prima cosa che voi avete cancellato. Mi auguro dal profondo del cuore, con grande rispetto per i colleghi della maggioranza e con ancora maggiore rispetto per i nostri figli, che non sia nei prossimi mesi il vostro primo rimpianto.

Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, signor Ministro, prima di intervenire sull'argomento della riforma dei Ministeri vorrei dire due parole

Ritornando sull'argomento, discutiamo oggi sull'opportunità di mettere insieme l'agricoltura e il turismo, che, tecnicamente, se vogliamo entrare nell'argomento, passa dai beni culturali al Ministero dell'agricoltura. Dal dibattito in Commissione è emerso evidentemente che non tutti siamo d'accordo, abbiamo appena sentito l'intervento del senatore Battistoni del Gruppo Forza Italia, che anche lui, con i suoi distinguo, non è d'accordo e il senatore Renzi, secondo il che effettivamente questa riforma non va. Credo però che bisogna guardare avanti, perché con questo provvedimento nasce invece un grande Ministero, un grande Ministero dell'agricoltura, un grande Ministero del turismo, che ci può dare grandissime

sappiamo tutti quanti, sono Patrimonio mondiale dell'Unesco - alla Valle dei Templi in Sicilia, c'è tutto un territorio da visitare, da ammirare, da apprezzare e da valorizzare. La gente viene volentieri in Italia, lo sappiamo, perché il nostro è effettivamente il Belpaese. A tutta questa gente, A tutta questa gente, a tutti questi turisti bisognerà pur dare ospitalità; a tutte queste persone bisognerà pur dare da mangiare e far apprezzare la nostra capacità consolidata: è una realtà consolidata il fatto che molti turisti scelgono molto spesso solo ed esclusivamente dei percorsi enogastronomici. È risaputo che, tra le altre cose, il nostro Paese è famoso in tutto il mondo

una parte importantissima della nostra capacità di fare agricoltura. Se poi vogliamo entrare nel dettaglio, abbiamo 4.700 tipicità regionali e questo ci fa capire la forza che la nostra agricoltura e i nostri agricoltori sono da sempre capaci di mettere in campo. È solo attraverso la valorizzazione e l'offerta capillare di tutta questa enorme biodiversità di prodotti che riusciremo a vincere la sfida della ricettività turistica: rispetto agli altri Paesi, la nostra agricoltura è un punto di forza per il settore enogastronomico. In questa direzione, valorizzando le piccole, ma buone produzioni dei nostri agricoltori, la Lega ha presentato un disegno di legge recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni locali». Lo abbiamo presentato proprio in questi giorni, in maniera tale da permettere agli agricoltori di vendere direttamente i loro prodotti, liberandosi così finalmente dalla morsa dei commercianti, che spesso e volentieri speculano sul prodotto

Il turismo enogastronomico e la ricettività collegata hanno potenzialità enormi. Pensiamo solo all'indotto dei *souvenir* alimentari: parlo dei prosciutti, dei salumi e dei formaggi. Queste sono le cose che i turisti vogliono portarsi a casa; è difficile portarsi a casa un mattone del Colosseo o un reperto storico - lo dico ovviamente con ironia - mentre un salume, un prosciutto o qualsiasi altro prodotto della nostra gastronomia i turisti lo portano a casa volentieri. È un indotto che sta crescendo in maniera enorme. Sappiamo che il settore degli agriturismi in questi ultimi anni sta crescendo di circa il 10 per cento annuo. Stiamo parlando di oltre

non solo per i prodotti riguardanti l'agricoltura ma anche per la ricettività balneare e per il settore ittico, rispetto al quale sicuramente abbiamo molto da dire. Cosa ci serve? Bisogna crederci e lavorare nella giusta direzione. Il riordino del Ministero dell'agricoltura e del turismo, di fatto, signor Presidente,

ministro Centinaio. Noi della Lega lo sosterremo sicuramente e convintamente. Buon lavoro, signor Ministro.

sottolineo: pare - senza aumento di costi a carico dello Stato. perché spesso i costi effettivi si misurano dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti, anche in termini di efficienza e sprechi, visto che molto spesso questi cambiamenti hanno conseguenze negative maggiori del previsto. Cosa diversa, invece, se andiamo ad analizzare il provvedimento sul piano politico. Faccio una considerazione di carattere generale, partendo dall'analisi dell'articolo 1, che prevede il trasferimento delle competenze sul turismo. A questo proposito non possiamo non sottolineare come il termine «cambiamento», tanto sbandierato dal MoVimento 5 Stelle, proprio alla luce di questo provvedimento, possa essere tradotto in stazionamento, invecchiamento. Chi volesse essere più romantico, potrebbe rinominarlo con il gattopardesco «cambiamo tutto perché nulla cambi»: nulla di diverso

è il testo scritto nel contratto di Governo, tanto sbandierato dal *leader* dei 5 Stelle, onorevole Di Maio, come la novità del secolo, un nuovo modo di fare politica, la grande svolta, che forse avete approcciato con troppa superficialità e vi ha portato subito Quindi, per ragioni di *Realpolitik*, si fa esattamente il contrario di quanto scritto. Colleghi, non ci scandalizziamo, ma semplicemente prendiamo atto della nuova situazione che si è creata, e speriamo che da oggi in avanti chi si erge a moralista lo faccia con più attenzione. Voglio comunque sottolineare che, rispetto a quanto enunciato nel contratto, riferendomi specificamente alla parte che vi ho appena citato e all'intero paragrafo relativo al turismo del contratto di Governo, Fratelli d'Italia ha un giudizio complessivamente positivo, perché le varie le varie proposte mirano a combattere la concorrenza sleale, gli abusi e le agenzie straniere che lucrano sul nostro patrimonio. Anche noi siamo favorevoli all'introduzione del Ministero del turismo. Oggi, però, discutiamo un provvedimento che nella sua parte iniziale vuole togliere al Ministero per i beni e le attività culturali

anche per un'idea generale del turismo legata fortemente al patrimonio artistico, archeologico e storico di cui il nostro Paese è ricco. se andiamo ad analizzare quanto sia complesso il sistema turistico nel suo insieme, scopriamo che il turismo culturale è uno dei tanti turismi che il nostro Paese può offrire e quindi non ci scandalizziamo né ci meravigliamo del fatto che ci sia un passaggio di competenze. Pensiamo, ad esempio, al turismo che ogni estate riempie le nostre spiagge di centinaia di migliaia di persone, dove di culturale - consentitemi consentitemi di dirlo - c'è ben poco, così come al turismo invernale che riempie le nostre montagne di appassionati di sci alpino; pensiamo al turismo termale e del benessere, dove, anche in questo caso, la componente culturale è molto scarsa.

Penso, in particolare, a tutti quei territori che non riescono ad intercettare il flusso turistico delle città d'arte, dove è concentrato il turismo culturale, ma che sono ricchi anch'essi di monumenti e tesori artistici, spesso spesso non conosciuti, e alle tante, tantissime sagre e manifestazioni locali, che hanno al centro i prodotti dell'agroalimentare italiano, che possono diventare meta di molti turisti. D'altra parte, andando indietro con la memoria, il turismo in Italia ha sempre avuto una vita travagliata; penso alla costituzione del Ministero nei primi anni Cinquanta, fino al *referendum* abrogativo, per poi tornare in auge come delega alla Presidenza del Consiglio, per poi passare sotto il Ministero delle attività produttive e poi

sul piano della pianificazione turistica, spesso demandata agli enti locali e spesso mal coordinata anche fra i vari enti territoriali. Penso che chi ha gestito fino ad oggi il Ministero per i beni e le attività culturali ha pensato poco alla pianificazione turistica nel suo complesso e ancor meno e e male a gestire il nostro patrimonio artistico e monumentale: penso ai nostri musei e siti archeologici. Sicuramente sarebbe stato meglio se avesse pensato a trovare più risorse per organizzare in modo migliore i nostri musei e a nominare meno direttori non italiani, come se da noi mancassero

di promuovere e valorizzare, in modo complementare, tutte le eccellenze del *made in Italy* espresse nei vari territori. Vedremo come saranno gestite le iniziative dei vari turismi, che hanno esigenze differenti, con criticità e problematiche specifiche e che necessitano di soluzioni altrettanto tuttavia ricchi di prodotti e opere, verranno valorizzati. Siamo convinti che il *made in Italy*, soprattutto quello agroalimentare, possa rappresentare una grande risorsa per la valorizzazione dei nostri territori. Pertanto, non valutiamo negativamente questo passaggio, anche se ribadiamo la nostra idea di un Ministero *ad hoc* per il turismo, ma lo facciamo con riserva, con la riserva di valutare il suo operato, signor Ministro: lo valuteremo con oggettività, senza pregiudiziali e nel merito, a seconda di come saprà valorizzare il comparto turistico nel suo insieme. Vorrei altresì evidenziare il nostro

e come questo provvedimento, con le disposizioni di cui all'articolo 3, inizi un percorso di sviluppo di questo Ministero. Abbiamo da sempre creduto che la famiglia sia la base della nostra società e che sia il il fondamentale e primario nucleo su cui si poggia l'intera Nazione. Ad oggi abbiamo visto, purtroppo da parte nostra, attuare politiche poco attente e spesso abbiamo visto in azione un pensiero culturale che mirava alla distruzione di questo istituto, dal *referendum* sul divorzio al riconoscimento Non voglio certo innescare un dibattito sul tema, ma sicuramente questo rappresenta un segnale forte di controtendenza. Non vorremmo, però, che questo fosse solo un Ministero di facciata e lo diciamo perché, a nostro avviso, mancano in questo progetto proposte concrete e incisive per dare un supporto vero alla famiglia. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo avanzato proposte: mi riferisco al fatto che gli asili nido siano non solo gratuiti, ma anche aperti fino all'orario di chiusura di negozi e uffici; vorremmo che fosse introdotto il reddito d'infanzia, con un assegno familiare di 400 euro al mese; vorremmo che si applicasse il quoziente familiare in ambito fiscale. Ma soprattutto vorremmo che si attuasse un vero e proprio piano di sostegno alla natalità e le proposte che noi offriamo a questo Governo e che ho appena elencato vanno in questa direzione. Noi abbiamo bisogno di far crescere il nostro Paese, la nostra

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il dibattito sul riordino dei Ministeri, nell'ottica del *made in Italy*, apre una questione squisitamente politica, che ci tocca tutti da vicino. Chi asserisce che la cultura non sia importante, che vada considerata a parte, chi ritiene che sia soltanto una fonte, di cui certe voci pesano troppo sul bilancio pubblico, evidentemente non ha compreso, né si è mai soffermato a riflettere su ciò che siamo noi, cittadini italiani, né tantomeno, nello specifico, come l'Italia debba la sua straordinaria importanza nel mondo alla cultura: la cultura rappresenta il nostro passato, la storia, la memoria, ma è anche il nostro futuro. La politica raramente pratica l'arte e la cultura, relegandole spesso e in modo sommario a mera finzione, a qualcosa di inutile, e considera gli artisti e gli intellettuali dei perditempo, non sapendo nulla della funzione profondamente etica dell'arte, soprattutto nella sua formidabile capacità di cogliere La cultura rappresenta ciò che è nel pensiero heideggeriano il linguaggio come casa dell'essere, dove «linguaggio» non può non significare anche essenza essenza o verità. Conosco abbastanza bene il mondo dei libri: non è, quella dei libri, una realtà fatta romanticamente di autori e storie, ma una vera industria, composta da *editor*, fiere, agenti, tutti protesi a creare quello che non è più soltanto cultura o bellezza, ma anche *business*. Questo è solo un esempio per determinare come debba essere compresa la necessità che vi siano Ministeri e persone di riferimento competenti, che conoscano il linguaggio della cultura e dell'arte e ne comprendano le esigenze, che riescano a interpretare la realtà della cultura come compenetrazione, intreccio tra idea, concetto e realtà e che non pensino che basti gestire le casse agli ingressi di musei, teatri o fiere. Possiamo mettere nelle mani di chiunque e staccare da una sinergia importante il futuro di enti che tutto il mondo ci invidia, come la Scala di Milano, l'Arena di Verona, il Maggio musicale fiorentino, il Festival di Spoleto? Rassegne cinematografiche, come la Mostra di Venezia? Imprese straordinarie, come il Salone il Salone del libro di Torino, che con Ernesto Ferrero è cresciuto sino a diventare un appuntamento di riferimento per l'editoria europea e non solo? Per non parlare della straordinaria qualità di un interminabile elenco di altre manifestazioni, che determinano l'essenza del nostro Paese e che va promosso in un contesto ampio e importante. Massimo Severo Giannini ha definito il cosiddetto bene culturale qualcosa che «offre testimonianza materiale avente valore di civiltà». Se cultura è civiltà allora è anche comunità. E qui potremmo fare riferimento al bene comune come bene che supera ogni esigenza individuale, come straordinariamente

spazio entro il quale si allarga il margine occupazionale. L'appiattimento di attività disgiunte tra loro a un unico comune denominatore può significare, quindi, una cosa soltanto: che stiamo omologando tutte le grandi eccellenze a un unico prodotto da *outlet*, segnato da un marchio di fabbrica quanto mai semplicistico. Ci sono manifestazioni pensate per il grande pubblico, ma non ci può essere vera ricerca senza spazi particolari di riflessione, adeguati a un uditorio più raccolto, diversamente consapevole o preparato. Attraverso questa ricerca verrà determinato lo spazio entro il quale la cultura italiana (e non solo, com'è ovvio) La cultura e la società sono strettamente connesse, costituiscono un insieme di saperi, costumi, comportamenti in cui ciascuno di noi come parte della stessa società si identifica. Franco Cardini nel 2017 definisce la cultura come «sapersi e volersi mettere in discussione», come «condizione di coraggio morale e intellettuale». «Desiderio di imparare, di ascoltare gli altri, di portare un contributo alla crescita». Auspico dunque che questo Governo e l'Italia facciano propria la consapevolezza che la cultura rimanga, come lo è stato nella scorsa legislatura, terreno di impresa e di diffusione creativa, di comunità, da definire in sinergia tra il Ministero della cultura, del turismo, su cui ha lavorato il ministro Franceschini, e quello dello sviluppo economico, per portare avanti un discorso di eccellenza che ci contraddistingue con il supporto delle singole Non sarà certamente casuale il fatto che tutti i regimi totalitari abbiano voluto mettere un bavaglio alla cultura: la mia comunità nazionale, quella slovena della Venezia Giulia, fu vittima di un vero e proprio tentativo di genocidio perpetrato durante il Ventennio fascista, con la soppressione di tutte le associazioni culturali, culturali, con roghi di case di cultura e di libri di biblioteche pubbliche e private, provocando un fuoriuscitismo in massa degli intellettuali sloveni, unico nell'Europa tra le due Guerre. Non vorrei che dovessimo richiamare le parole di Alcide de Gasperi, che nel 1913 parla - lo cito - «di una parabola discendente della nostra Non è decadenza la volontà di far convergere problematiche e necessità in un calderone che ha più il sapore di un *franchising* che non di Ministeri con delle serie basi programmatiche che è la politica a dover indicare? Non le sembra pericoloso, signor Presidente, onorevoli senatori, pensare che stiamo scivolando verso un *finis terrae*, dando il segnale alle generazioni future come non ci si debba preoccupare dell'educazione al pensiero critico *tout court*? Saremo in grado di tollerare generazioni future, convinte che la rete o le immagini condivise sui vari *social* determinino o rappresentino la verità e la realtà assolute? È una politica culturale seria, congiunta a una politica sulle sue possibilità di sviluppo, a dover dare ai giovani gli strumenti per valutare criticamente ciò che apprendono. dicendo che, nella consapevolezza dell'unicità e dell'inestimabile valore del patrimonio culturale italiano, bisogna creare delle sinergie serie per svilupparlo, prendere coscienza che la cultura riguarda ciascuno di noi in prima persona, e che è la politica a doverne portare la responsabilità,

nello specifico il provvedimento che trasferisce le funzioni in materia di turismo fino ad oggi esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'attribuzione al Ministro per la famiglia e le disabilità delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità. Un provvedimento che nel suo complesso se, da una parte, va nella direzione dell'ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane ed economiche, dall'altra tende a tende a connettere e ad armonizzare materie e settori che non è più pensabile di trattare a comparti stagni e in modo separato. Rispondo alla senatrice Malpezzi, che si stupisce di fronte a un provvedimento davanti al quale io, invece, mi sarei aspettata di vedere l'approvazione e l'appoggio di chi era al Governo nella passata legislatura e oggi si trova ai banchi dell'opposizione, e proprio dai miei colleghi è stato fortemente criticato mettendo in evidenza una grande contraddizione della loro politica. È stato criticato il fatto che in questo riordino il turismo sia stata ricompreso all'interno del Ministero dell'agricoltura, adducendo come motivo principale il fatto che esso abbia registrato negli ultimi anni una crescita, al contrario dell'agricoltura, e che in tal modo si rischia di farlo retrocedere. Mi sembra, cari colleghi, che sia una motivazione molto fragile, che non tiene conto di quanto il turismo, che finora è stato in capo al MIBACT, abbia giovato dell'attività

gli ex Ministri dell'agricoltura e del turismo andavano a braccetto, e proprio l'ex Ministro del turismo - al turismo, lo sottolineo - aveva elaborato un programma che prevedeva che, dopo l'anno dei cammini e dei borghi, il 2018 sarebbe stato l'anno del cibo, con l'obiettivo di avviare manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica dell'Italia. Tutto questo per dire che chi oggi siede ai banchi dell'opposizione sa benissimo che il turismo ha bisogno dell'agricoltura, perché non si può di esso parlare senza abbinarlo al cibo, il quale a sua volta ci riporta all'agricoltura, a quella tradizione contadina che da secoli ha curato le nostre terre, portando come frutto le materie prime che sono alla base dei nostri prodotti tipici,

cosa varrebbe visitare Parma, la mia bella città, senza assaggiarne il prosciutto, il parmigiano o senza visitarne le bellissime campagne e colline che la circondano. Nella mia piccola esperienza nel settore turistico mi sono assolutamente convinta che il turismo abbia bisogno dell'agricoltura e che quest'ultima sia un traino importante per il turismo. Lo dicono anche i pacchetti turistici che vengono confezionati dalle più importanti aziende di *marketing* turistico. Chiedo ancora se siete davvero convinti che il florido turismo toscano sarebbe stato tale senza le distese di girasoli delle sue colline e i suoi ordinati vigneti e uliveti. Il turismo ha bisogno dell'agricoltura e questo lo dimostrano anche le infinite sagre che da decenni si svolgono nei nostri paesi, nei nostri piccoli Comuni italiani che in quelle occasioni, proprio proponendo i prodotti tipici del territorio, registrano flussi di turismo che diversamente non ci sarebbero. Solo per fare un esempio, una piccola frazione del parmense di soli 58 abitanti con la sua storica sagra della polenta è capace di attirare fino a 10.000 persone ogni anno. un esempio fra tanti, che i miei colleghi in Parlamento che sono anche sindaci, consiglieri o assessori possono confermare, riconoscendo l'importanza di eventi del genere, che altro non sono che feste dei frutti della terra. Castelli ne abbiamo e chiese altrettanto, ma cosa mi può portare a scegliere dì visitarne uno piuttosto che un altro? È chiaro che la scelta dipende non solo dalla loro bellezza, ma anche dal contesto paesaggistico in cui sono inseriti, dalle tradizioni, dalla cucina, dal cibo del luogo in cui si trovano. E ancora, per ultimo voglio ricordare come il turismo definito una volta di nicchia stia sempre

se non quella di avere un unico Ministero che se ne occupa, mettendone in relazione le reciproche caratteristiche? Non è questo - come affermano molti - il capriccio di un Ministro. Anzi, colgo l'occasione per augurare al ministro Centinaio un buon lavoro. È un modo nuovo per stare al passo con le esigenze e le aspettative dei turisti. Il turismo ha fame, il turismo ha bisogno dell'agricoltura e questo è il messaggio che con il provvedimento in esame vogliamo far passare. Sarei stata ben contenta se su questa partita che interessa l'economia italiana ci fossimo trovati tutti d'accordo. Al G20 l'hanno capito che agricoltura e turismo stanno insieme, tanto che il documento è stato votato all'unanimità. Concludo con un breve cenno relativo al Ministero della famiglia e della disabilità, ricordando a tutti che la disabilità è un qualcosa che prima di tutto va chiamata col suo nome, con profondo rispetto, e che i problemi della disabilità non possono essere trattati in modo staccato dalla materia famiglia.

Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 definisce - a nostro avviso - «riordino delle attribuzioni dei Ministeri» un riequilibrio politico interno al Governo, sbagliato anche se politicamente legittimo e distante, molto distante, dalle concrete reali esigenze dell'Italia e dei Ministeri oggetto del presunto riordino. Voi che narrate il cambiamento imponete, con la decretazione d'urgenza, la restaurazione del manuale Cencelli: due Ministeri al ministro Di Maio richiedevano un rafforzamento del Ministero dell'agricoltura per il ministro Centinaio. Noi rimaniamo convinti di un utilizzo forzato dell'uso della decretazione. Lo abbiamo spiegato abbondantemente e molto bene nella pregiudiziale che abbiamo discusso in questa sede. Ovviamente, io sostituirei la parola «riordino» con la parola «pasticcio», perché è la confusione, più che la ragione, che guida i concetti essenziali degli articoli di legge oggetti del presente decreto: quattro articoli che si presentano privi di un comune denominatore; privi di una visione di Governo; privi di una riflessione sul versante delle politiche da attuare nei diversi Ministeri e privi - e questa è la cosa ancor più grave di un'analisi delle risorse necessarie per attuare nuove politiche per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Al contrario, ci si occupa dell'equilibrio delle poltrone. Colleghi senatori, la narrazione vola, il Governo latita, così come latita l'attuazione del vostro contratto di Governo. All'articolo 1, infatti, la scelta di spostare il turismo dall'attuale Ministero dei beni culturali al Ministero delle politiche agricole non ha una immediata evidenza nelle relazioni e nel rispetto di ciò che il turismo rappresenta per il prodotto interno lordo del nostro Paese, oltre il 12 Si fa demagogia pensando a una relazione naturale che esiste tra il turismo e il sistema dell'agroalimentare, dei nostri giacimenti enogastronomici, che però in realtà rappresentano poco più del 5-7 per cento dell'intero PIL che il comparto turistico rappresenta. Se si vuole investire nel turismo, una piattaforma naturale come l'Italia richiede nella riduzione delle distanze, nella connessione tra le diverse infrastrutture aeroportuali

Volendo fare una scelta razionale, tutto ci porta a pensare che il turismo dovrà sempre di più rappresentare un perno fondamentale dello sviluppo economico e sociale del Paese. È agricoltura, certamente, ma è anche innovazione, Industria 4.0, *made in Italy,* moda, Motor valley*,* il frutto dell'attrattività economica di un Paese, straordinariamente importante sul piano culturale come l'Italia; una piattaforma culturale naturale,

sarà e rappresenterà un danno importante e pesante per il Paese. Quando la vostra narrazione terminerà e ci si misurerà sugli aspetti fondamentali del Governo, si scoprirà che le strutture di missione avevano obiettivi precisi, alcuni dei quali peraltro già avviati: il rilancio degli investimenti; il rimettere al centro la prevenzione del nostro fragile, ma bel Paese; la realizzazione di un grande piano piano nazionale di cura, di rammendo e di rigenerazione della nostra Italia. Le strutture di missione avevano rappresentato anche l'occasione per ristabilire una relazione più proficua tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Non è vero che si saturavano e si demolivano le relazioni con il comparto delle autonomie locali. In questi anni, anche grazie alle scelte che abbiamo attuato, eliminando il patto di stabilità, i primi importanti segnali sulla ripresa degli investimenti erano stati attuati e le strutture di missione avevano rappresentato nella scuola, come nel recupero della prevenzione e del dissesto idrogeologico, un punto di riferimento essenziale. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Penso che giungerà il momento nel quale noi dovremo fare una riflessione seria, della quale la narrazione dovrà lasciare spazio all'azione concreta di governo. Presidente, questi sono gli aspetti più importanti. Giudichiamo negativamente proprio perché privo di qualsiasi azione concreta per lo sviluppo economico e sociale, per la crescita dell'occupazione e del lavoro. di riordino delle funzioni all'interno di Ministeri, l'obiettivo fondamentale del Paese dovrebbero essere la crescita economica, il rilancio dell'occupazione e soprattutto l'investimento sull'identità fondamentale che l'Italia ha a disposizione, che sono gli italiani, la loro creatività e la loro capacità di agire. La vostra narrazione continua invece a dare come punto di riferimento il «ci pensiamo noi», con la solidarietà più che con la sussidiarietà, negando diritti fondamentali che richiedono un investimento delle risorse umane. L'Italia è un grande Paese, ecco perché la vostra narrazione impatterà negativamente sull'Italia che crede in un futuro migliore.

quindi evidente che si parla di una provvisorietà; e noi sappiamo che in Italia tutti i provvedimenti, quando sono provvisori, poi di fatto diventano definitivi. Quindi, bisogna essere molto coraggiosi nel poterli prospettare in modo definitivo. Chiedo allora un coraggio particolare ai 5 Stelle e agli amici della Lega, nonché al Presidente della Commissione e al Ministro, per fare in modo che, posto che l'agricoltura è un comparto fondamentale e merita tutta l'attenzione possibile, alla pari il turismo, che è la prima industria del nostro Paese, abbia organizzazione, fondi, personale e possibilità di prossimità. E vi dico ciò perché l'ho sperimentato sulla mia pelle, essendo stata commissaria dell'Azienda autonoma di turismo dell'isola di Capri, la perla del mondo. Quando parliamo di turismo, Capri è la nostra perla in Italia.

Presidente, colleghe e colleghi, il nostro Gruppo voterà contro il provvedimento in esame e nella dichiarazione di voto integreremo una serie di motivazioni. Io vorrei parlare solo del turismo e fare alcune osservazioni. Ho sentito le motivazioni per cui si è deciso, da parte del Governo, di portare il turismo all'agricoltura. Si dice che il turismo ha bisogno di agricoltura. Sì, il turismo ha bisogno di agricoltura e di enogastronomia. Il turismo, però, ha bisogno anche di infrastrutture; il turismo ha bisogno di servizi; il turismo ha bisogno di qualità nella sanità; il turismo ha bisogno di tutto, perché è uno di quei fattori fondamentali per lo sviluppo che integra le politiche. Ciò di cui non ha bisogno il turismo

Di che cosa avrebbe bisogno il turismo? Prima di tutto - a mio parere - ha bisogno di un progetto, di un progetto integrato, che metta al centro le priorità del turismo. Ne ho sentito parlare poco. La prima priorità è l'organizzazione: siamo un Paese indietro di vent'anni rispetto all'organizzazione turistica.

Bisogna adeguare le nostre strutture ricettive con un progetto di investimenti capace di sostenere anche un'impresa piccola, che ha poche camere e una capacità di rilancio

E questo non lo possono fare né un Ministero, né le Regioni. È indispensabile costruire un progetto di promo-commercializzazione che metta al centro gli operatori

Ma l'organizzazione e la strategia qui non vedo. Vedo piuttosto il tentativo di costruire un equilibrio di potere, che è pienamente legittimo.

riorganizziamo i rapporti e le relazioni con le Regioni e scegliamo i mercati strategici su cui costruire la nostra promo-commercializzazione. Diamo un nuovo ruolo agli operatori che debbono costruire reti capaci di stare sui mercati

di aggregare domanda, organizzarla in modo da portare valore aggiunto, perché i numeri non bastano. Dobbiamo collegarci a sistemi di medio-alto valore aggiunto Grazie,

Lei ha la delega e sa bene con quanta debolezza la porta a casa dal punto di vista della struttura del Dipartimento. C'è da riorganizzare l'ENIT.

realizzi un progetto, metta attorno a un tavolo i diversi protagonisti e ricostruiamo una rete capace di stare nel mondo. Noi non abbiamo il problema di dire che l'Italia è bella. Lo sanno tutti; basta guardare tutte le indagini a livello mondiale: siamo sempre ai primissimi posti nell'immaginario dei cinesi o degli indiani. Il problema è che non abbiamo gli strumenti per rendere

piccola, subalterna alla visione secondo cui il turismo ha bisogno di agricoltura. Il turismo ha bisogno di tutto: ha bisogno di un progetto e di una cultura industriale, che purtroppo nella proposta che fate davvero non vedo.

l'impianto normativo del provvedimento in esame nel complesso prevede norme sicuramente condivisibili, sebbene - come ho avuto modo di dire già durante la discussione della questione pregiudiziale - avremmo apprezzato la presentazione di un disegno di legge e non l'utilizzo della decretazione d'urgenza, considerata, anche in questo caso, non necessaria. necessaria. L'impianto normativo dispone di cinque articoli. Se da un lato, incide su fattori fondamentali per l'economia nazionale (in particolare, quelli del turismo o dell'ambiente), con uno spostamento di competenze e di prerogative che avrebbero, a tal fine, richiesto, proprio per siffatti motivi, un maggior tempo nella valutazione delle norme; dall'altro lato, dovrebbe, almeno teoricamente, favorire un processo di velocizzazione decisionale determinato dall'accorpamento di funzioni e deliberazioni in capo a un singolo Ministero su specifiche tematiche rispetto a quanto avviene proprio oggi. Certamente, come tutte le leggi, ogni impianto normativo può essere perfettibile e suscettibile di miglioramenti. Bisogna quindi attendere - questo è il nostro auspicio l'impatto che le disposizioni previste dal decreto-legge avranno sul tessuto sociale ed economico del Paese per poter dare un giudizio più incisivo e certo sull'efficacia di queste norme. Tuttavia, non può essere ritenuto un ordinario passaggio di competenze il riordino di alcuni Ministeri, considerato come si incide in modo significativo sulla *governance* - ad esempio - delle emergenze ambientali, di azione di prevenzione e sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio, a partire proprio da quello scolastico. inoltre, su un comparto strategico per la nostra economia, il turismo. Con il passaggio delle competenze al Ministero delle politiche agricole, che trova la nostra piena condivisione, si valorizza il turismo italiano anche attraverso la produzione agroalimentare, al fine di avviare una politica integrata di valorizzazione del *made in Italy*. Sul trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'ambiente per gli interventi di emergenza ambientale, volti a garantire la sicurezza agroalimentare del territorio della Regione Campania, della Regione Campania, abbiamo invece fortissime riserve. Non è chiaro - ad esempio - se, nell'ambito delle misure di ordine di competenze e attribuzioni di nuovi compiti, il Ministero dell'ambiente avrà anche quello di gestire un capitolo così difficile Grazie, è assolutamente necessario fare chiarezza affinché la struttura nazionale della Protezione civile e le strutture regionali di supporto abbiano il massimo appoggio da parte delle istituzioni nell'ambito della definizione di un quadro normativo certo e chiaro. desidero aggiungere che è importante creare una grande sinergia tra tutte le istituzioni locali, provinciali e regionali. Pertanto, a mio avviso, siamo di fronte a un decreto-legge che presenta sicuramente delle luci, ma anche tantissime ombre. In relazione agli interventi attribuiti al Ministero delegato per la famiglia e la disabilità in materia di coordinamento delle politiche di tutela dei diritti della famiglia, per l'infanzia e l'adolescenza e in favore delle persone con grande disabilità, anche con riferimento all'inclusione scolastica, all'accessibilità e alla mobilità, non possiamo non sottacere che gli stanziamenti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità sono nettamente insufficienti rispetto alle effettive esigenze che necessitano anche oggi. Auspichiamo a tal fine, pertanto, che in occasione della prossima legge di bilancio il Ministro competente possa prevedere adeguati fondi in favore della disabilità. disabilità. Apprezziamo invece a tal fine l'interesse del ministro Fontana giunto in corsa sull'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze. Siamo di fronte a un decreto-legge che, accanto a misure che trovano il nostro consenso - penso ad esempio alla norma approvata in Commissione, che consente di siglare un protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute per la definizione delle misure sanitarie per il contrasto al diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze - ne contiene altre che invece non ci convincono. Avete soppresso la struttura di missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, Casa Italia - come qualcuno ha ricordato prima - tutte strutture che sicuramente consentivano trasparenza e

Sulla struttura di missione, che aveva una sorta di gestione nella procedura relativa ai fondi derivati dallo sblocco del patto di stabilità per i Comuni, non è chiaro - ad esempio - chi svolgerà l'azione di monitoraggio sullo stato di attuazione per gli interventi sulle verifiche di vulnerabilità sismica, le cui competenze passeranno nel fondo unico dell'edilizia scolastica, in capo al Ministero dell'istruzione. Un'analisi più approfondita delle norme sarebbe stata sicuramente auspicabile. L'auspicio è che il passaggio di competenze e di prerogative tra i Ministeri interessati possa rafforzare e migliorare il sistema-Paese, per le materie che sono state coinvolte dal decreto-legge. Da parte mia, non potrà che esserci la massima

e le imprese derivanti dall'accorpamento delle funzioni dei Dicasteri coinvolti. In caso contrario, attraverso le prerogative derivanti dalla funzione di parlamentare, insieme ai miei colleghi di Fratelli d'Italia sarò pronto nelle Aule del Senato a correggere eventuali distorsioni derivanti dall'applicazione delle norme

che mi trovano particolarmente e totalmente in disaccordo. Al fondo di questa mia inquietudine, che cercherò di spiegare più avanti, c'è la scelta della maggioranza di istituire un Ministero della famiglia e della disabilità. Oggi, nel 2018, la famiglia, questa nostra grandissima e bella istituzione affettiva e sociale, è molto fragile ed è forte nello stesso tempo, di fronte alle intemperie e agli accidenti, dal lavoro dei giovani, alla perdita del lavoro delle madri e dei padri, alle separazioni, alla difficoltà degli adolescenti, al rapporto scuola-famiglia. La famiglia si sostiene solo attraverso l'emancipazione delle persone che la compongono, a partire dalla condizione delle donne. In questo senso, andava recuperata la storia istituzionale del nostro Paese, con i Ministeri delle pari opportunità. Questo avrebbe dovuto essere di insegnamento per proseguire un percorso avviato vent'anni fa. Non si torna indietro, relegando le problematiche a un Ministero per la famiglia e le disabilità dimostrando una concezione arretrata della società. La famiglia sta bene se sta bene la società e viceversa; sta bene se c'è un sistema di *welfare* che l'accompagna. Non condivido, quindi, la scelta di sottrarre sottrarre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - come hanno detto anche molto bene i colleghi che mi hanno preceduta - e competenze riguardo, in particolare, al sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e quelle relative al coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il tema per la nostra società, il tema di tutti, riguarda l'emancipazione sociale ed economica: si tratta di aumentare l'occupazione femminile e fare in modo che le donne non lascino il lavoro La maternità è un valore sociale e come tale va incoraggiata e sostenuta. Trovo poco lungimirante chi pensa di sostenere e conciliare l'attività lavorativa con le responsabilità derivanti dall'educazione e dall'accudimento dei propri figli istituendo un Ministero della famiglia. Lavoro e famiglia vanno tenuti insieme ed è per questo che ritengo che questo tema vada affrontato in armonia con le politiche pubbliche di *welfare*, da una parte, e con la contrattazione, dall'altra. Questa *ratio* - ad esempio - è stata seguita per lo stanziamento nel 2017 e nel 2018 di circa 110 milioni di euro di sgravi contributivi per il sostegno alla contrattazione di secondo livello, per misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e lavoratrici innovative e migliorative. Che facciamo? Stacchiamo questo insieme di provvedimenti e lo isoliamo in un Ministero? Per quanto riguarda il trasferimento delle politiche in favore delle persone con disabilità, faccio due esempi: la bellissima legge della scorsa legislatura sul «Dopo di noi» e quella sui *caregiver*. La legge sul dopo di noi è nata per accompagnare le famiglie: solo chi non ha mai parlato con una famiglia, con un genitore, con una madre e un padre che devono rimanere sereni quando non saranno più in grado di accudire i propri figlioli, non sa quanto lavoro di accompagnamento Non sa quanto lavoro delicato va fatto, perché i genitori possono portare le loro preoccupazioni fuori dalle mura familiari e affidarsi a una rete di servizi sociali. La famiglia deve affidarsi a una politica pubblica, altrimenti non ce la fa. Quanto è grande Quanto è grande il lavoro di contatto umano che svolgono i nostri assistenti sociali. Quanto è grande il lavoro delle associazioni di terzo settore. Per questo non si può spezzettare la competenza sul dopo di noi tra due Ministeri, con doppie firme. Non eravate quelli della semplificazione? Proprio un anno fa, nel luglio del 2017, è stato approvato il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, che si fonda sul principio di uguaglianza sostanziale per persone con disabilità per rispondere alla giusta e ineludibile richiesta di cittadinanza piena e integrale delle persone con disabilità, in coerenza con le previsioni e la Convenzione ONU sui loro diritti. Ebbene, la promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione sono da considerare non più settori dell'intervento di *welfare*, quanto piuttosto criteri ispiratori complessivi per tutti, anche per le persone che sono meno deboli. Per questo motivo ribadisco la coerenza nel lasciare la competenza della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto riguarda, infine, la scelta al bilancio della Presidenza del Consiglio la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei *caregiver* familiari, al termine della scorsa legislatura è stato fatto un grandissimo lavoro *bipartisan* per ottenere questo fondo. Non è stato facile: il Parlamento è stato impegnato grandemente su questo

nell'attività bella e delicata di cura - come avviene già in tante esperienze regionali - e considerati beneficiari di politiche trasversali. Quindi, Presidente - e Quindi, Presidente - e chiudo - sono molto preoccupata di questo arretramento. Spero che nel Paese insorga una risposta di pressione sociale molto forte. Non vorrei che dovessimo avere come spettro quel bellissimo quadro di Goya dal titolo «Il sonno della ragione genera mostri». Io sono però molto fiduciosa e in questo tempo in cui si dice che non c'è più differenza tra centrodestra e centrosinistra

per la libertà di una famiglia che ha una persona con disabilità di poter affidare il proprio figliolo a una

*(PD)*. Un Ministero per la famiglia e la disabilità isola, non apre. Noi vogliamo accompagnare il sogno di libertà ed emancipazione dei nostri concittadini e delle loro famiglie. I tempi sono duri, ma ce la faremo. l'impressione di avere tagliato il suo intervento nella parte che sembrava fosse quella finale. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ci troviamo ad affrontare provvedimenti di notevole importanza per rendere ancora più efficace l'operato del Governo e per ottenere risultati concreti, a miglioramento della vita dei cittadini del nostro Paese. Mi riferisco ovviamente al trasferimento delle competenze sul turismo al Ministero delle politiche agricole, nonché all'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia in tutte le sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine precipuo del contrasto alla crisi demografica. In Italia stiamo assistendo a una sempre più accentuata crisi delle nascite: secondo i dati ISTAT, nel 2017 si è registrato un nuovo *record* negativo, minimo storico dall'unità d'Italia. Illustri economisti e demografi confermano il nesso tra crisi della natalità e andamento dell'economia. Le politiche in favore della famiglia sinora adottate non sembrano, dunque, essersi rivelate efficaci ai fini del superamento della crisi demografica. Serve una programmazione strategica delle politiche familiari, una regia più ampia e complessiva dell'azione di Governo, capace di indirizzare e promuovere in modo sinergico le diverse politiche volte al sostegno e al benessere della famiglia e al rilancio della natalità, dando impulso a interventi selettivi in ogni ambito, *in primis*, quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura. Ecco il perché di questo provvedimento, che ci trova totalmente favorevoli, per un cambio di registro e per una maggiore attenzione nei riguardi delle politiche per la famiglia e per lo sviluppo della natalità, con conseguente crescita del nostro Paese.

Mi permetto pertanto di consigliare alle opposizioni un'attenta lettura dell'articolo 29 della nostra Carta costituzionale, dove viene sancita a chiare lettere l'unicità della famiglia e la sua distinzione rispetto alle altre formazioni sociali, che vengono riconosciute e regolate altrove. Chi non è d'accordo può sempre promuovere una proposta di riforma costituzionale e della legge naturale cui la Carta costituzionale rimanda. Per quanto concerne agricoltura e turismo, sono entrambi elementi fondamentali per il tessuto economico, produttivo e sociale del nostro Paese: due categorie di eccellenza dell'Italia di cui andiamo orgogliosi, invidiate ed emulate in tutto il mondo. Oggi, con il provvedimento che andiamo a discutere, si intende trasferire questo messaggio non solo all'opinione pubblica, ma anche e soprattutto nella geografia dei Ministeri. Personalmente condivido questo riordino, che nobilita due grandi eccellenze del nostro Paese, come appunto turismo e agricoltura. Chi, come il sottoscritto, proviene da una terra a forte vocazione turistica e agricola, come la Liguria, non può che accogliere con favore ed entusiasmo questa scelta. Mi permettano e mi perdonino, signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, una piccola parentesi personale. Io nasco, appunto, in terra ligure, nella provincia di Savona in particolare, e sono cresciuto a Laigueglia, piccolo borgo marinaro affacciato sul mare, per cui, ogni singolo momento della mia infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta l'ho trascorso a stretto contatto con il turismo e l'agricoltura e tutto ciò che rappresentano questi settori, ricchi di straordinarie potenzialità, il tutto incastonato in una meravigliosa terra come la nostra Italia, la quale ha una predisposizione unica per essere vocata al turismo: è contornata dal mare e impreziosita dalle isole, protetta dalle montagne, riempita da colline e pianure, colma di storia e tradizioni. Il turismo è un po' come un libro: non dipende dallo scaffale in cui è riposto, gentilissima senatrice Malpezzi, ma dai suoi contenuti, da ciò che ha da offrire, dalle emozioni che trasmette leggendolo, se ti incuriosisce, se ti fa riflettere e - perché no - se ti fa sognare. Un po' come quando avete sognato di vincere il *referendum,* lo ricorda? Per questo, signor Presidente, ammetto di trovare poco produttiva la discussione su dove collocare le deleghe che fanno riferimento al turismo e bene fa il ministro Centinaio

in discussione rappresenta un'occasione senza precedenti: promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari

cui si indica il turismo come mezzo di promozione dei territori e strumento atto a sviluppare ulteriormente l'agricoltura, essendo una attività di reddito supplettiva per gli imprenditori agricoli. Bravo, Ministro! Del resto, il Ministro durante la sua relazione ha affermato con chiarezza che il turismo è un settore industriale ad alta incidenza imprenditoriale, fondamentale per la nostra economia (il 13 per

«In virtù della concessione e i concessionari demaniali possiedono suolo e strutture, quindi la concessione è un bene, non è un servizio». Qualcuno può pensare che i piccoli miglioramenti di questi ultimi tempi siano il frutto di un'oculata gestione, ma non si può non tenere conto di quanto il mondo sia diventato molto poco accogliente in questi ultimi tempi e che il nostro Paese per i turisti, soprattutto quelli italiani, era forse l'unico modo per potersi regalare un po' di vacanza. Spero sia finito il tempo degli improbabili *spot* di promozione in un inglese tentennante, di portali *web* lanciati in grande stile e poi finiti nel dimenticatoio, di strutture nazionali che non incrementano la competitività, anzi. Con questa innovazione organizzativa sarà finalmente possibile valorizzare la produzione agroalimentare attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, dando l'opportunità a chi visita l'Italia di conoscere il nostro Paese anche attraverso le produzioni tipiche, creando finalmente un *brand* nazionale una sinergia mirata ad affiancare settori (turismo e agricoltura, in senso lato, comprensivo di tutti i settori di attività inclusi in tale concetto) indubbiamente trainanti per l'economia italiana, promozione del territorio e la tutela delle tradizioni. L'innovazione del settore turismo non passa dalla sua collocazione, ma dipende da altri fattori. Positive sono l'intenzione e l'intuizione del Ministro dell'interazione con gli altri Ministeri, con i quali operare in sinergia e facendo gioco di squadra.

e lo so bene), della connessione (è l'era digitale) e di molto altro. Alla luce di tutto questo, la certezza per noi è che questa scelta rappresenta un'opportunità per un decisivo cambio di passo verso un'ulteriore valorizzazione di turismo, agricoltura, *made in Italy* ed eccellenze italiane. Questo Questo è il Governo del cambiamento, anche di mentalità. Anche attraverso questo tipo di iniziative si evince un messaggio chiaro, anzi, Ministro, chiarissimo in questo senso: il turismo al centro dell'agenda del Governo è un grande, grande segnale di cambiamento. Grazie, Ministro, grazie, Governo!

Signor Presidente, signori Ministri del Governo, onorevoli colleghi senatori,

questa relazione biunivoca tra l'agricoltura - l'enogastronomia, per valorizzare l'Anno nazionale del cibo, che è appunto il 2018 - e il turismo è l'inizio di una riforma più ambiziosa, va bene; non siamo d'accordo, ma aspettiamo che lei faccia questa riforma più ambiziosa. Quindi, riprendendo solo la conclusione del mio discorso (che diventerebbe il terzo, quindi sarebbe un po' noioso), lei non dimentichi che l'industria del turismo è la più digitale in assoluto e quindi pensi a questo Dipartimento del turismo e all'agenda digitale. Infatti, i flussi turistici internazionali devono essere studiati in termini di *big data*

2, relativo al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente, visto anche il programma di Governo che il ministro Costa ci è venuto a illustrare in Commissione (la lotta ai cambiamenti climatici, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, la salvaguardia della natura, la valorizzazione dell'acqua, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, lo sviluppo dell'economia circolare e la politica dei rifiuti zero: questi erano i sei o il Ministro, circa un mese fa è venuto a raccontarci in Commissione), ci saremmo aspettati, con maggior coraggio, l'istituzione di un nuovo Comitato interministeriale - presieduto certamente dal Ministro dell'ambiente - vista la strategicità e la centralità

riveste certamente una centralità importante. L'attuale Comitato, ascrivibile solo alla Regione Campania e sorto nel 2013 per evidenti ragioni di urgenza, avrebbe dovuto completare, dal 2013 al 2018, le sue funzioni. Quindi, in maniera più ambiziosa, un nuovo Comitato interministeriale presieduto dal Ministro dell'ambiente, centrale rispetto a una serie di altri Ministeri, sarebbe stato certamente un segno di cambiamento e di maggiore coraggio. Passo, poi, all'articolo 3, che riguarda la famiglia.

con riferimento a questi tre grandi argomenti (mondo femminile, natalità e famiglia, che non sono mai stati affrontati in maniera organica, come se fossero secondari rispetto a tutta una serie di altri temi che riguardano maggiormente lo sviluppo economico) ci saremmo aspettati che questo Governo li avesse affrontati all'interno di un'agenda di trasformazioni economiche, sociali, culturali e industriali che che permeasse l'impresa, la famiglia e il terzo settore. per esempio, alla valorizzazione del mondo femminile, un mondo estremamente organizzato, con qualità specifiche, che sono veramente adattabili al terzo settore. Bene, tutto ciò non è avvenuto. Perché diciamo questo? Perché, hanno detto anche dei colleghi che mi hanno preceduto, dobbiamo analizzare brevemente alcuni dati che ci devono assolutamente preoccupare. Sappiamo che l'Italia è il Paese europeo con il minor tasso di fecondità e occupazione femminile. E le tendenze del futuro non sono certamente incoraggianti. I dati ci dicono che da circa quarant'anni i tassi di fecondità sono molto bassi e l'indicatore (meno di due figli per ogni donna) è assolutamente inferiore a quanto sarebbe richiesto per garantire il semplice ricambio generazionale, con evidenti ripercussioni negative sia sulla sostenibilità del sistema pensionistico e fiscale, ma anche sulle prospettive di crescita del sistema economico. L'Italia, inoltre, è il Paese più anziano al mondo, dopo il Giappone, e anche questo ci deve far riflettere. Ci saranno 74 over per ogni 100 attivi (e per attivi intendo le persone tra i venti e i sessantaquattro anni), a fronte degli attuali 38. Questo succederà non tanto lontano, nel 2050. I nuovi nati sono diminuiti drammaticamente. Vi do alcuni dati. Nel 1916 erano 676.000, nel 1945 821.000, nel 1965, l'anno del *boom* economico, 1,35 milioni, nel 2016 sono scesi drammaticamente a 474.000. Questi dati vanno analizzati con riferimento anche a delle indagini socio-economiche che sono state fatte. Abbiamo dei dati, riferiti a campioni molto diversificati, che dicono che la volontà di costruire una famiglia in Italia è molto alta:

per cento si fermerebbe ad un figlio e solo il 6 per cento non ne vorrebbe. Quindi, questi sono dati che ci devono far riflettere, proprio per costruire delle politiche che vadano incontro alla volontà e ai desideri di questi ragazzi. Sappiamo anche che, tra le famiglie che hanno tre o più figli, l'incidenza della povertà assoluta aumenta quasi del 50 per cento, passando dal 18 per di carattere più economico, che riguarda la produttività. Non perché voglia dire che la produttività può aumentare se coinvolgiamo maggiormente le donne oltre che attuando politiche fiscali sul costo del lavoro di maggiore attenzione verso gli imprenditori per evidenziare che la produttività in Italia nel 2018 cresce solo dello 0,6 per cento, a fronte dell'1,2 della Francia e dell'1,3 della Germania, proprio perché il mondo femminile è meno

che, nel 1999, disse che il Giappone era in declino perché non lasciava spazio alle donne. Koizumi, che era Primo ministro nel periodo 2001-2006, ruppe con la tradizione adottando delle misure concrete per incoraggiare la partecipazione e la valorizzazione del mondo femminile nel mercato del lavoro. Le donne, per intenderci, iniziavano ad essere decisamente più frustrate e erano anche meno feconde. Questo è stato provato scientificamente. Non possiamo dire che il nuovo millennio sia iniziato per il Giappone con dati positivi solo per questa ragione, certamente, però il collegamento tra il maggior coinvolgimento del mondo femminile e la crescita economica del Giappone ci dovrebbe far riflettere. Mi avvio a concludere. Costruiamo attorno a

donne; non politiche di genere come «la Ministra», «la sindaca» e cose di questo tipo, ma una politica di valorizzazione delle qualità del mondo femminile che sono completamente diverse da quelle del mondo maschile. Il mondo femminile è molto più organizzato, più altruistico, più empatico, più sensibile, maggiore comprensione per tutte le problematiche sociali ed anche maggiore capacità organizzativa. È un mondo che bisognerebbe coinvolgere maggiormente, attraverso la tecnologia, nei processi organizzativi che servono a migliorare la nostra economia, perché il modo di ragionare delle donne è decisamente diverso da quello degli uomini: è un modo di ragionare molto più orientato all'organizzazione e alla capacità di fare tante cose insieme

Tratterò alcuni aspetti che mi coinvolgono anche come professore di geofisica. Il provvedimento trasferisce dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'ambiente le funzioni in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo. Si sopprime la struttura di missione ItaliaSicura contro il dissesto idrogeologico e non viene rinnovato il mandato della struttura di missione ItaliaSicura scuole per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Il Dipartimento Casa Italia diventa un progetto gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Immagino che tali strutture furono pensate per tre ordini di motivi: pericolosità sismica ed idrogeologica del territorio italiano; grande vulnerabilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture; paurosi ritardi nelle politiche di prevenzione dei grandi rischi, che da sempre ci fanno vivere in continua e drammatica emergenza. La nostra è una penisola con grandi pericoli naturali, a causa della complessa geofisica del sottosuolo e della natura geologica, che ci rendono tra i Paesi più sismici e più franosi del mondo. Il dissesto si intreccia con una grave carenza nella pianificazione del territorio. La regola base della prevenzione strutturale non è stata quasi mai rispettata. Dal 1950 ad oggi contiamo circa 5.500 vittime in oltre 4.000 tra frane e alluvioni, oltre che danni plurimiliardari. Franano anche strade e autostrade, ferrovie, reti idriche ed elettriche. Inoltre, oggi rileviamo un'ulteriore accelerazione del dissesto idrogeologico, a causa dei cambiamenti climatici innescati dal surriscaldamento globale. Il deterioramento del territorio è un pesante aggravio nei conti dello Stato e accumula debito futuro. Anche in una visione strettamente ragionieristica, è utile investire in prevenzione; è un investimento a grande moltiplicatore. Per il rischio sismico, annotiamo mediamente un terremoto di intensità maggiore o eguale all'ottavo grado della scala Mercalli ogni quattro anni e mezzo. Dal 1968 (terremoto della valle del Belice), in cinquant'anni ci sono stati dieci severi scuotimenti, con danni per 150 miliardi di euro e drammatiche conseguenze, economicamente non valutabili, in termini di vite umane, di disgregazione sociale e di perdita o danneggiamento del patrimonio culturale. In Italia, l'alta pericolosità associata alla vulnerabilità del costruito e all'esposizione della popolazione, determina un rischio critico. Emblematica la situazione delle scuole per il rischio sismico: l'esposizione è massima e la vulnerabilità elevata. Su 42.000 edifici scolastici solo 13.000 sono successivi all'entrata in vigore della prima seria normativa antisismica del 1976. Oltre il 40 per cento degli edifici scolastici si trova in zona 1 e 2, cioè interessate rispettivamente da terremoti fortissimi e forti; meno del 15 per cento di tali edifici è progettato o adeguato con criteri antisismici sufficienti. Sulla base dell'elevato e ben noto rischio idrogeologico e sismico, possiamo affidarci a strutture di missione? Non sono queste strutture straordinarie, emergenziali? Concentrare i poteri e/o commissariare i problemi va bene per eventualità eccezionali ma in condizioni di persistente cronicità, come nel nostro caso, è un grave errore. I nostri rischi naturali hanno una normale gravità e vanno gestiti da strutture ministeriali e territoriali finalizzate a ciò, adeguatamente potenziate e finanziate. In particolare, il Ministero dell'ambiente, da un ruolo marginale nella difesa del suolo e mitigazione dei rischi, deve assurgere a un ruolo primario. Il persistere di strutture di missione ci farebbe tornare indietro di trentadue anni a quando il Ministero dell'ambiente non esisteva ancora. Inoltre, che senso ha regimentare i corsi d'acqua ma continuare a consumare suolo? Che senso ha contenere le frane ma non contrastare adeguatamente gli incendi boschivi dei versanti? La prevenzione va operata da monte a valle in modo organico e in ciò solo il Ministero dell'ambiente può avere un quadro unitario.

Non si può condividere la passata prassi, fin troppo abusata, di non far funzionare l'ordinario per costringerci allo straordinario. Non possiamo continuare ad essere la patria dell'emergenza, con le ignobili risate alle tre di notte del 6 aprile 2009 mentre giovani innocenti spiravano sotto le macerie della Casa dello studente a L'Aquila. Terremoti, frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche sono i violenti, normali, fenomeni naturali dell'Italia, tra l'altro abbastanza conosciuti da noi studiosi e in buona parte abbastanza prevedibili. Diventano catastrofi per gravi colpe umane. I 27 angioletti del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel sisma del 2002 pesano sulla coscienza della politica. Quel paese era «NC», sismicamente non classificato secondo la normativa allora vigente e quindi non assoggettato a criteri antisismici, mentre da cinque anni esisteva una nuova classificazione sismica, lasciata ad impolverarsi nei cassetti, che lo poneva in seconda categoria per la quale necessitano severe strutture antisismiche, capaci di resistere a terremoti ben più forti di quello che ha sbriciolato la scuola. Odo il grido di dolore di tutte le vittime delle cosiddette catastrofi naturali. Prevenzione! Per il rischio sismico è indispensabile una specifica microzonazione sismica, una valutazione di vulnerabilità e un adeguamento di tutto il costruito. Per il dissesto idrogeologico vanno eliminate le cause scatenanti, valutati i guasti prodotti ed eseguiti gli interventi di bonifica. Se non dovesse essere possibile ottenere la messa in sicurezza del costruito, si potranno attuare opportune delocalizzazioni. In tutto ciò, solo il pieno funzionamento del Ministero dell'ambiente può garantire il successo. Ma per intervenire occorre una valida e aggiornata cartografia tematica (e qui casca l'asino). La nuova carta geologica d'Italia copre solo il 40 per cento del territorio nazionale; mancano molte aree ad elevatissima pericolosità sismica ed idraulica, come ad esempio quasi l'intera Calabria. Inoltre, la gran parte delle Regioni non ha un ufficio geologico. Anche la professionalità geologica è fortemente sottovalutata. Da tutto ciò scaturisce la necessità di creare strutture normali di gestione del territorio e dei rischi, atte ad affrontare il necessario studio, la bonifica, la tutela e la valorizzazione degli strepitosi beni ambientali e socioculturali italiani. Occorre quindi dotare strutturalmente il Ministero dell'ambiente perché possa intraprendere una lotta integrata al degrado fisico e antropico del territorio, con finanziamenti ancor più consistenti di quelli elargiti alle strutture di missione, ma spesi in modo più sapiente e con le dovute priorità d'intervento. Occorre un cambio di paradigma nella visione politica: l'ambiente non deve essere più lo squallido recapito di processi insostenibili, ma il punto di partenza per costruire uno sviluppo ecosostenibile e duraturo. L'ambiente prima di tutto; per una vita dignitosa e non solo per una mera sopravvivenza.

Signor Presidente, ho ascoltato con attenzioni tutti gli interventi; spenderò poche parole sulle questioni relative al turismo e alla famiglia perché vorrei poi concentrarmi sulle altre. Per quanto riguarda il turismo, mi sembra del tutto evidente e chiaro che non si tratta di abbandonare delle esperienze, delle sinergie positive e delle attività svolte all'interno del MIBACT per promuovere unitariamente la cultura e il turismo. Si tratta di aggiungere altre sinergie; si tratta di trovare nuove opportunità di crescita, anche in termini di nuovi posti di lavoro. Quindi l'ambizione è semplicemente quella di affrontare una visione di sistema adeguata alle esigenze e alle potenzialità di più settori; una cosa non esclude assolutamente l'altra. Quindi non solo le attività agricole e agroalimentari, ma anche il patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e anche l'offerta delle strutture ricettive. Per quanto riguarda la famiglia, la scelta di rendere più coerente la disciplina si è resa necessaria per la profonda crisi delle nascite, come alcuni di noi hanno già sottolineato. Nel 2017 abbiamo raggiunto il picco massimo di questa crisi con la nascita e la registrazione agli uffici comunali del minor numero di bambini dall'inizio della storia del nostro Paese fino ad oggi. È evidente che i Governi precedenti hanno fatto troppo poco per tutelare la famiglia. Le politiche adottate sono state del tutto insufficienti per superare la crisi demografica e i fatti ne sono la testimonianza diretta. Il Governo del cambiamento darà quindi impulso ad interventi in ogni ambito, economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura, per fermare la crisi demografica e rilanciare la famiglia una volta per tutte. Fino ad oggi anche la disabilità è stata gestita in modo molto frammentato con competenze sparse all'interno di vari Ministeri. Da ora in avanti la Presidenza del Consiglio sarà la sede propria per dare il giusto impulso alle politiche in favore delle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità. quindi ai temi che mi stanno più a cuore, che sono quelli relativi alle competenze del Ministro dell'ambiente, del Ministro delle infrastrutture e in particolar modo alla soppressione di di ItaliaSicura e di Casa Italia, di cui il presidente Renzi ha fatto una strenua difesa fino a poco tempo fa. Il Governo intende cancellare strutture che rappresentano delle duplicazioni di costi per la finanza pubblica e occuparsi di prevenzione di rischio idrogeologico e sismico in maniera strutturale e sistematica con le vie ordinarie. Questo è il nostro intento. Nella passata legislatura abbiamo visto nascere diverse strutture presso la Presidenza del consiglio, chissà, forse frutto di una diffidenza del Presidente del consiglio *pro tempore* nei confronti dei propri Ministri. Quel che è certo è che l'accentramento dei compiti in capo al Presidente del Consiglio ricorda molto da vicino la logica del «*ghe pensi mi*» di berlusconiana memoria; un «*ghe pensi mi*» in salsa fiorentina, verrebbe da dire. La logica dell'uomo solo al comando che risolve i problemi è una logica che ha accomunato destra e sinistra e che in realtà non ha mai risolto nessun problema nel nostro Paese; questa logica non ci apparterrà mai. Nello specifico, Casa Italia ha prodotto risultati decisamente inferiori alle aspettative e anche durante le audizioni non è mancato chi lo ha fatto presente. Per esempio, il presidente del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati ha dichiarato che i territori e i cittadini non hanno compreso quale fosse la missione di questo ente. Anche il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri non ha usato mezzi termini, dicendo che sul tema della prevenzione del rischio sismico Casa Italia non ha operato, ma si è prodotto solo un documento di scarsissimo impatto dal punto di vista della prevenzione sismica. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e la chiusura di ItaliaSicura, noi vogliamo ridare centralità al Ministero dell'ambiente su un tema che da sempre è stato di sua competenza, individuando nel Ministero un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per le azioni di contrasto al dissesto. Il ministro Costa ha già assicurato pubblicamente che il contrasto al dissesto idrogeologico sarà una delle priorità del suo Dicastero e intende attivarsi per sbloccare i fondi e fornire supporto alla progettazione degli interventi prioritari. Però occorre dire una cosa molto chiara: il dissesto idrogeologico si combatte, prima di ogni altra cosa, con una seria e rigorosa legge contro il consumo di suolo, che ovviamente i precedenti Governi si sono ben guardati dall'approvare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Si è parlato molto e a sproposito delle opinioni degli auditi in Commissione, come ho già citato all'inizio. Sono state espresse molte richieste di chiarimento, ma è naturale che sia così, di fronte a un cambio organizzativo come quello in questione. Tuttavia nessuno ha gridato allo scandalo nei confronti di questa scelta organizzativa; anzi, qualcuno ha esplicitamente criticato l'esperienza di ItaliaSicura, come il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha dichiarato che la struttura di missione ItaliaSicura non è stata in grado di fare coordinamento con gli enti, utilizzando in maniera coerente e più rapida le risorse.

In effetti, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle strutture idriche ha il suo punto di forza unicamente nella pubblicità e nella comunicazione. È servita a fare grandi annunci e a presentare *slide* in giro per l'Italia in convegni appositamente organizzati e sempre sponsorizzati da Palazzo Chigi.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, ItaliaSicura ha realizzato il cosiddetto portale dell'acqua; c'è un'interessante rassegna di norme e di dati statistici editi da Istat e una mappa interattiva, dalla quale si evince lo stato drammatico della depurazione in Italia e il numero impressionante di procedure di infrazione. Per superare l'emergenza, il CIPE nel 2012 ha stanziato 1,6 miliardi di euro per 183 interventi di collettamento e di depurazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Ad attuare tale intervento è stato chiamato un commissario straordinario, che ha fornito assistenza dal 2013 al 2015 al Ministero dell'ambiente. L'attività della struttura di missione su questo tema non ci pare per nulla rilevante. Anche per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, abbiamo un'apposita sezione del sito di ItaliaSicura con una rassegna di norme statistiche e di dati tratti dai rapporti di ISPRA, infarcita di centinaia di *spot* propagandistici per raccontare e riraccontare le cose fatte da altri, allietati da gioiosi *selfie* delle maestranze impegnate nei cantieri, attivi indipendentemente dall'attività della struttura di missione. Prendiamo ad esempio il cavallo di battaglia della struttura di missione, il Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, e il recupero del cosiddetto tesoretto di 2 miliardi di euro non spesi negli anni precedenti. Enunciato così, il Piano nazionale di opere e di interventi di riduzione del rischio idrogeologico parrebbe un piano organico risolutivo, sostenuto da un progetto unico e da un programma economico. In realtà, si tratta di un piano che comprende un elenco di interventi inseriti dalle Regioni in una piattaforma digitale sviluppata e gestita dall'ISPRA per conto del Ministero dell'ambiente ancor prima dell'istituzione della struttura di missione. Andiamo ad analizzare il tesoretto dei 2 miliardi recuperati, secondo ItaliaSicura, dalla revoca dei finanziamenti e dagli interventi finanziati dal Ministero prima del 2010 e mai realizzati. Ebbene, grazie a un'interrogazione della scorsa legislatura della nostra deputata Federica Daga abbiamo saputo che il recupero del reale non ha raggiunto i 7 milioni di euro: altro che 2 miliardi. miliardi. Anche questo era uno dei soliti annunci della struttura di missione, naturalmente ripreso con enfasi dai giornali. In conclusione, il Ministero potrà tranquillamente continuare a fare il lavoro che ha sempre fatto prima, durante e dopo la struttura di missione, senza sentirne alcuna mancanza. finestra"). Avverto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, una proposta di non passaggio all'esame degli articoli da parte del senatore Ferrari. La votazione sarà effettuata dopo le repliche della relatrice di minoranza e del rappresentante del Governo, prima dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1

di essere alleati del Partito Democratico - hanno detto in quella sede. Ho ascoltato con grande interesse il dibattito qui in Aula e anche la cortesia dei toni utilizzati dal collega Vallardi, che indubbiamente ha una grande esperienza come sindaco, e volevo dispiacermi con lui, perché in Italia, nel corso degli ultimi tre anni e mezzo, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, sono stati 12.415 gli interventi e 8.114 gli edifici coinvolti e se nessuno di questi interventi ha riguardato i Comuni da lui amministrati mi dispiace. Ci sono invece tanti sindaci,

stanno sollevando perplessità e preoccupazioni perché non sanno a chi rivolgersi ora. Siccome questa è la prerogativa che il Governo dovrebbe avere, ossia rispondere ai cittadini, la prima domanda che abbiamo provato a fare è stata proprio questa: se le competenze passano al MIUR, ci sarà un semplicissimo numero numero di telefono che consentirà agli amministratori locali, che - lo ribadisco - non hanno colore, di fare quel numero e trovare qualcuno che risponda, impedendo loro magari di fare errori nella programmazione e nella progettazione, come spesso è accaduto negli anni precedenti? *(Applausi dal il problema non riguarda chi smonta e chi costruisce, chi fa, chi mette e chi toglie; il problema è se i soldi che ci sono arrivano a chi poi deve utilizzarli per il bene dei cittadini. E le strutture di missione servivano a questo:

che non sia necessario ascoltarli che stiano dicendo chissà cosa, prendendo le posizioni di chi governava prima, mi sembra quantomeno assurdo. Provo ad andare con ordine. Lo dico alla collega Saponara, che ha fatto un intervento assolutamente interessante rispetto al turismo e alla scelta che - saremo sciocchi noi - non riusciamo ancora a capire. Cara collega Saponara, lo dico sempre attraverso il Presidente - non è che voi unite semplicemente il turismo all'agricoltura, ma che vi dimenticate completamente in questo modo che si chiama turismo culturale e che comprende anche

Per voi si ragiona per compartimenti stagni, quasi per ghetti e devono essere quelli. Non sapete neanche cosa sia la sinergia tra le diverse forze che operano tra loro. Turismo culturale:

Ripamonti, che ha fatto un intervento indubbiamente complesso. Con coraggio, se volevate valorizzare il turismo, non potevate creare il Ministero del turismo da solo? Potevate fare una scelta molto più chiara e più trasparente. Sarebbe stata semplicissima. Lo avreste valorizzato in tutti gli aspetti, senza dover passare del tempo a spiegare una scelta che oggettivamente è immotivata da qualsiasi punto di vista. vista. Caro senatore Ripamonti, sempre tramite la cortesia del Presidente, aggiungo che lei ha affrontato nel suo intervento anche la tematica delle politiche familiari dicendo, come veniva ribadito anche poco fa, che l'Italia sta subendo e vivendo il grandissimo crollo delle nascite, un grandissimo calo demografico e che, quindi, è necessario attuare delle politiche per la famiglia.

un coordinatore (di che?) che vada ulteriormente a burocratizzare un sistema che, invece, deve essere semplificato con politiche che siano davvero attive. E che si ragioni davvero sulla composizione oggi - a lei non piacerà - delle famiglie perché la mia famiglia è diversa dalla sua ed è diversa da quella di qualcun altro. Non piacerà a lei, ma si guardi in giro; non c'è una famiglia uguale all'altra. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Le può piacere o meno, ma le famiglie, fortunatamente, sono diverse. Fortunatamente - dico io - il mondo in cui viviamo è un altro. Aggiungo ancora un'ultima questione, che per me è importante. Lo abbiamo ribadito più volte all'interno di quest'Assemblea e siamo anche stati un po' simpaticamente

Noi abbiamo una convinzione chiara: turismo e cultura - su questo vogliamo che voi ci smentiate - sono gli elementi distintivi del *brand* Italia e il nostro Paese è al primo posto davvero nel *ranking* mondiale della *brand* *reputation*. In questo senso è necessario approcciarsi in un altro

come anticipato, passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, in base all'articolo 96 del Regolamento.

molti interventi che hanno contestato il passaggio delle competenze in materia di turismo al Ministero dell'agricoltura con tesi diverse, tutte molto interessanti nel merito, partendo da chi sosteneva l'utilità di lasciare le cose come stanno a chi affermava l'opportunità di trasferire la competenza al Ministero per lo sviluppo economico; altri hanno chiesto la costituzione di un Ministero apposito, alcuni hanno addirittura chiesto che la competenza sul turismo passasse alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono tutte soluzioni che devo dire, senza nemmeno una grande necessità di approfondimento, apparivano subito molto superiori alla soluzione che invece è stata scelta dal Governo, con il passaggio delle competenze al Ministero dell'agricoltura. Devo dire che questa è sembrata subito - l'ha detto poco fa il senatore Errani - una scelta molto piccola, una scelta, cioè, senza nessun tipo di prospettiva. Peraltro, anche chi ha sostenuto in Commissione e in Assemblea, anche poco fa, l'utilità del passaggio al Ministero dell'agricoltura lo ha fatto con argomenti - devo dire - molto deboli. Oggi pomeriggio in Aula ho

Le ragioni di questo spostamento sono due e sono note a tutti noi. C'è innanzitutto l'omaggio - debbo dire, dal punto di vista di chi lo fa, anche meritato - al senatore Centinaio, La questione si è combinata evidentemente con con i risultati del bilancino dei poteri tra i due partiti che sostengono il Governo, e nel bilancino dei poteri ci stava che il turismo venisse spostato da un Ministero all'altro. Queste sono le due ragioni per le quali il Governo propone questo spostamento. Io credo che per ragioni di questa natura si possano fare molte cose: vediamo che addirittura si possono nominare i consiglieri delle Ferrovie dello Stato,

cosa molto molto diversa: lo spostamento di competenze per motivi di parte politica è una cosa che noi finora non avevamo mai visto. Io dico questo e mi

noi evitiamo di esercitarli per seguire un'indicazione politica sbagliata.

Grazie, Presidente,

Ci sono due urgenze per far fronte in maniera adeguata al dissesto idrogeologico e a tutte le altre questioni afferenti allo stesso, di cui stiamo parlando da alcune ore oggi in questa La prima è superare la frammentazione dei poteri, che purtroppo ha determinato l'inefficacia di moltissimi interventi che erano pur nati sotto i migliori auspici. L'altra cosa da fare è lavorare superando la straordinarietà degli interventi, concentrandosi in particolare sulla questione della prevenzione. Ovviamente, accanto a questo, c'è la necessità degli investimenti. Orbene, la frammentazione era esattamente il motivo per cui i Governi precedenti hanno costituito le unità di missione, di cui molto si è parlato in questa sede. La questione centrale, signor Presidente, sta nel fatto che c'è bisogno di una *governance* unitaria per superare la frammentazione, e la *governance* unitaria è l'unico modo per realizzare davvero una politica, una *policy* generale davvero efficace ed efficiente. La *ratio* per cui era stata inserita sotto la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi di grandi personalità - è stato citato prima l'architetto Renzo Piano, ma potremmo citarne anche altri - stava esattamente in questo ragionamento. Mi riferisco cioè alla capacità di una struttura snella, capace di coordinare gli interventi, di essere efficace, di superare la frammentazione, capace di essere credibile, di essere unico interlocutore con gli enti locali, coi Comuni, con le Città metropolitane, con le Province, con le Regioni e con tutti gli enti nazionali e territoriali di cui la nostra Nazione non manca.

Pensiamo forse che questi 14 enti di monitoraggio avranno una riduzione dal punto di vista dell'azione del Governo, oppure

pregiudizialmente interventi migliorativi che possono sempre essere fatti. È del tutto evidente che quando si affrontano attività di Governo, tutte le azioni e le decisioni devono essere messe in discussione, valutando i punti di forza e i punti di debolezza, ma in questo caso, come già diceva il presidente Zanda, la vera motivazione di questo provvedimento - e anche la discussione odierna lo fa emergere in maniera evidente - è una spartizione dei poteri che prescinde totalmente dalla finalità dell'efficienza e dell'efficacia per i cittadini, ma risponde invece - questa sì - a una logica neospartitoria da manuale Cencelli. È evidente che questi sono i motivi per cui noi abbiamo proposto l'emendamento 2.1; un emendamento draconiano che non vuole difendere lo *status quo,* ma

di indire dei concorsi presso il Ministero dell'ambiente, c'è una reale esigenza. Spero che, dopo il trasferimento in pianta stabile, strutturale, all'interno del Ministero dell'ambiente, si affronti una volta per tutte

3.10 per il quale chiediamo una riformulazione. Con esattezza,

sulla questione, che è stata affrontata in vari interventi che mi hanno preceduto, riguardante il singolare nella intitolazione e nel testo dell'articolo 3, riguardante la famiglia. In realtà, forti trasformazioni sociali intervenute negli ultimi decenni hanno fortemente modificato la struttura, il ruolo, la fisonomia della famiglia. Oggi noi ci troviamo di fronte a una costellazione e a una pluralità di famiglie. Quindi, non possiamo più parlare al singolare. Non è solo una questione grammaticale. Lo stesso regolamento del censimento, il regolamento anagrafico e i dati ISTAT ci dicono che la famiglia modale classica è ridotta a poco più del 30 per cento, a fronte invece di una pluralità di modelli di famiglia che comprendono le famiglie ricostituite in seconda unione, le famiglie monogenitoriali, le famiglie monopersonali, adottive, affidatarie. Credo quindi che continuare a parlare di famiglia al singolare sia lesivo della pluralità, sia inopportuno rispetto al nostro tempo e sia anche offensivo nei confronti di quei bambini che si trovano all'interno di queste famiglie diverse, alcuni dei quali sono discriminati anche dalle parole del ministro Fontana, il quale ha affermato che non si possono riconoscere i figli di coppie dello stesso sesso. Ci piaccia o meno, questi bambini non hanno scelto in quale famiglia nascere, quindi hanno diritto a essere destinatari di cura, di attenzione educativa da parte dei loro genitori in qualsiasi contesto.

senatori Grassi

di Renzo Piano, senatore a vita e grande architetto ma non solo, anche di scienziati di chiara fama del calibro del professor Azzone, all'epoca rettore del Politecnico di Milano. È stato ricordato oggi che nella scorsa legislatura facemmo sul tema un dibattito di livello su una relazione, appunto, di Renzo Piano, cui parteciparono con grande condivisione tutti i Gruppi. Ma che cos'è, o dovrei dire purtroppo che cos'era il progetto Essenzialmente il passaggio dalla cultura dell'emergenza ad una cultura della prevenzione, intervenendo sul patrimonio immobiliare. Ho sentito che anche senatori della maggioranza insistevano su questo tema. Il patrimonio italiano è tanto bello quanto a rischio, nei centri storici, e a volte molto meno bello, se non brutto, ma altrettanto insicuro nelle periferie costruite negli anni Sessanta. Uno straordinario progetto studiato per la sicurezza degli italiani…

alla lettera *a*) premettere la seguente: "*0a*) *all'articolo 1, comma 8, sostituire le parole*: «Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo

la cancellazione di Casa Italia, come Partito Democratico, ritenevamo opportuno e necessario che i progetti relativi al rapporto sulla promozione della sicurezza dei rischi naturali, il progetto dieci cantieri e la mappa dei rischi naturali fossero da mantenere, anche in capo alla Presidenza del Consiglio. In realtà, da quello che si capisce, la maggioranza vuole cancellare tutto. Come non esprimere allora preoccupazione, dal momento che non c'è solo il declassamento, ma anche la cancellazione vera e propria di un'esperienza che noi reputiamo positiva, anche perché innovativa rispetto al passato?

UV))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, annuncio il voto di astensione del Gruppo Per le Autonomie al decreto-legge n. 86 sul riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Con riguardo al turismo, secondo noi non è rilevante a che Ministero aggregarlo, ai beni culturali piuttosto che al MISE, piuttosto che all'ambiente, piuttosto che all'agricoltura. Ovviamente, per l'importanza che il turismo ha per questo Paese, noi avremmo anche visto un Ministero a sé: ciò darebbe importanza a questo strategico settore della politica italiana. [**Presidenza

Se pensiamo alle bellezze, alle città di Roma, Venezia o Firenze, alle tantissime città d'arte, ai borghi medievali, alle varietà del paesaggio, alle montagne più belle del mondo, le Dolomiti, alle maestose vette delle Alpi occidentali, alle colline, al mare stupendo, alla cucina italiana, al *made in Italy*, alla creatività degli italiani, veramente l'Italia avrebbe il potenziale e dovrebbe essere il numero uno come meta turistica al mondo,

però è importante dare professionalità a questo Ministero. Se adesso un operatore del turismo è a capo di questo Ministero, io spero che porti in questa materia la sua professionalità e la sua esperienza. Ciò serve veramente, perché bisogna confezionare bene i tantissimi prodotti turistici; il Ministero avrà da compiere un intenso e a volte anche difficile lavoro di coordinamento. Però nel turismo non c'è bisogno di una strategia *top down*, bensì di una strategia *bottom up*, ossia di valorizzare e coordinare le tantissime offerte e i tantissimi prodotti turistici delle tantissime destinazioni d'Italia. Il Ministero non dovrà imporre, ma piuttosto avrà il compito di proporre, di agevolare, di incentivare e soprattutto di organizzare il turismo. È stato detto che ci vuole l'organizzazione del turismo e delle proposte Grazie, più che il Ministero, più che la politica. Sono loro che alla fine fanno i prodotti o non li fanno bene. Gli italiani per buona parte fanno bene il loro lavoro, ma ci vuole ancora più professionalità e ci vuole soprattutto l'aiuto da parte di un Governo che veda il turismo come obiettivo principale di una strategia politica per il Paese.

ma voglio dire al signor Ministro soprattutto una cosa: non è solo la politica turistica che fa il turismo, ma ci vuole anche un'efficiente politica per le infrastrutture, un'efficiente politica per la mobilità ci vuole anche sicurezza in tutto il Paese, perché il turista viene solo dove si sente sicuro e si sente bene. Ci vogliono quindi strategie politiche che non riguardino solo il turismo; queste sono importantissime per il turismo,

l'ho ricordato poco fa - di sopprimere alcune strutture di missione e portare le competenze, come nel caso della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, all'interno del Ministero competente. Grazie,

perché nel momento stesso in cui si dà vita a un Ministero della famiglia e della disabilità si fa, a nostro avviso, un'operazione pericolosa

perché può dar vita a operazioni di ghettizzazione: questo è il problema che è davanti a noi. Ovviamente, spero che questo non accada.

del decreto dignità. Invece, qui si fa solo e unicamente un'operazione ideologica, sotto il segno, ancora una volta, della Lega, che è il partito - Presidente, lei sarà molto contento - che dà l'impronta

la costruzione di un progetto nazionale in un settore che dovrebbe essere il *core business* del nostro Paese. Ebbene, ancora una volta, la scelta operata con questo decreto-legge di staccarlo dal Ministero dei beni culturali

certamente basato sui beni culturali del nostro Paese (abbiamo il 60 per cento dei beni culturali del mondo, ci mancherebbe altro!), così come le nostre risorse enogastronomiche sono fondamentali, le risorse ambientali lo sono altrettanto (il turismo ambientale, anch'esso, costituisce un nuovo percorso

all'interno del Ministero dell'ambiente, perché siamo convinti che riportarli in modo strutturale all'interno di Ministeri va bene. Non ci piace però, assolutamente, l'idea che, ancora una volta, possa essere soltanto una questione di sistemazione all'interno dei Ministeri. Su questo bisogna investire,

non lo facciate e che prendiate le distanze - le dichiarazioni che hanno accompagnato e che continuano ad accompagnare questo benedetto Ministero neocreato. Per tutti questi motivi, proprio per le scelte sbagliate in particolare su questo Ministero, che sono - ripeto

Signor Presidente, colleghi, io mi devo scusare con questa Assemblea e con la Presidenza per il mio comportamento inadeguato avuto qualche tempo fa col senatore Laus. Permettetemi però di spiegare perché ho avuto quel comportamento inadeguato. Laus, fino a poco tempo fa, gestiva una cooperativa di offerta di lavoro di multiservizi, quindi per lavoratori esternalizzati, diciamo, e li pagava - e li paga tuttora - tra i 3,50, i 4 e i 5 euro.

regionale, i suoi lavoratori e chiese chi non volesse abbassarsi lo stipendio. I lavoratori che alzarono la mano furono licenziati. Fu poi condannato dalla corte d'appello, quarta sezione penale di Torino,

Sta intervenendo per fatto personale, quindi io lo faccio parlare per il tempo che necessita di parlare, non sta insultando nessuno. Posso dirigere io l'Aula, scusate? Prego senatore. AIROLA *(M5S)*. Sto motivando la mia ira di quel giorno. Uno di quei lavoratori, Altieri, licenziato ingiustamente e poi, appunto, riconosciuto ingiustamente licenziato, lavorava al museo del cinema e scrisse a Ken Loach, regista che da anni si occupa di problemi di lavoratori, che quell'anno non venne a ritirare il premio speciale per lui. Quel premio rimase lì fino a quando non si sarebbe risolto questo problema. questo problema. Anche oggi che Laus ha lasciato la Rear in mano a congiunti (moglie e marito) i lavoratori continuano a essere pagati 3,50 euro. Quello che voglio dire è che quando lo incontrai tempo fa (era ancora consigliere), Laus mi disse che era la legge che gli permetteva di pagare così poco; gli risposi che anche nell'Ottocento in Virginia si poteva avere un campo di lavoratori gratis, ma che io non l'avrei fatto perché è una questione morale, non di mercato e si possono pagare 9 euro, cioè il prezzo giusto, i lavoratori anche senza bisogno di una legge.

senatore Laus, per fatto personale. Io spero che non diventi un dibattito fra senatori. Si rivolga comunque alla Presidenza ed ha tre minuti; così come tutti gli altri senatori. LAUS *(PD)*. Presidente, io devo ringraziare il senatore Airola - ma lo dico dal profondo del cuore - perché mi mette e ci mette nelle condizioni di entrare nel cuore di un problema.

di mettere in condizione imprenditori come Laus di non retribuire legittimamente, con contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più rappresentative, con una retribuzione oraria lorda che è anche - ahimè - di 5 euro. Queste sono le motivazioni che inducono il senatore Laus e altri colleghi a finalmente una legge che preveda il salario minimo orario, perché ci sono circa 3 milioni di lavoratori che non riescono a percepire un reddito decoroso e dignitoso. Ieri c'era il Partito Democratico: e dite che ha sbagliato. Oggi ci siete voi, ci sono i colleghi

casa un lavoratore che ha posto in essere comportamenti decisamente riprovevoli. Il giudice ha ritenuto che ci fosse un'ingiusta causa e il lavoratore è stato risarcito. Volevo ringraziare il senatore Airola per le scuse, ma probabilmente non conosce bene il significato, né dell'educazione, né delle scuse.

Signor Presidente, la notizia della morte del caporal maggiore De Mattia ha lasciato la città di Angri, e non solo, nello sgomento più profondo. Certo, quando un ragazzo di venticinque anni decide di togliersi la vita, è la società tutta a doversi interrogare sul perché e su cosa non è stato fatto affinché questo episodio così angoscioso e terribile non si verificasse. Enrico De Mattia, cittadino di Angri, proveniente dal 1° Reggimento granatieri di Sardegna, inquadrato nell'operazione Strade sicure, sabato scorso ha posto fine alla sua vita utilizzando la pistola di ordinanza mentre era in servizio presso Palazzo Grazioli. Grazioli. Sulla morte di Enrico va però fatta chiarezza, con la massima attenzione possibile. L'episodio deve essere approfondito in quanto si tratta del terzo suicidio in sei mesi di un militare impegnato nell'operazione Strade sicure. I militari ingaggiati in questa operazione seguono uno speciale *iter* addestrativo teorico e pratico, tale da garantire una pronta risposta operativa alle varie situazioni e sempre adeguata alle circostanze. Vista la delicatezza del tema, sarebbe necessario però mettere in campo un opportuno sistema di monitoraggio dello stato psicologico di tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate per affrontare il disturbo da *stress* cronico che - ahinoi - troppo spesso genera la scelta orribile del suicidio. Lo Stato deve sostenere i suoi militari, promuovendo percorsi di sostegno e supporto psicologico agli uomini delle Forze Armate. Enrico era un militare pieno di vita, un nostro conterraneo che, purtroppo, ha deciso di farla finita. Per ogni giovane vita che perdiamo, un pezzo di speranza di un futuro migliore se ne va. Esorto chiunque viva con difficoltà la vita a rivolgersi ai propri cari e giammai ad abbandonarsi a tragiche soluzioni. Oggi in quest'Assemblea desidero esprimere, anche a nome di tutto il Movimento,

Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, è mio dovere intervenire adesso, in questa Assemblea, alla fine dei lavori, come cittadino, come medico, come rappresentante delle istituzioni e Capogruppo di Forza Italia nella Commissione igiene e sanità del Senato, per far per far presente all'Assemblea quanto di grave sta accadendo in queste settimane all'ospedale metropolitano di Reggio Calabria, in particolar modo al Pronto Soccorso.

- per la quale ho chiesto al ministro Grillo, giovedì scorso, di mettere la parola fine al commissariamento. Mi auguro che, quando riceverò la sua risposta, il Ministro possa finalmente comunicare al sottoscritto e a tutti i calabresi la fine di un commissariamento che dura da undici anni. Da molto tempo i pazienti che arrivano al Pronto Soccorso di Reggio Calabria con fratture, lussazioni e distorsioni vengono stabilizzati con pezzi di cartone. Per chi non avesse sentito sono pronto a ripeterlo tutta la serata, tutta la notte: il problema è che oggi in Calabria il soccorso per chi ha una frattura viene prestato con pezzi di cartone. È quanto denunciato poche ore fa dal «Corriere della Calabria». Succede di notte, quando il reparto di ortopedia è chiuso a causa della carenza di personale che opera soltanto dalle ore 8 alle ore come se la sera, dalle ore 20 fino alle ore 8, tutti diventiamo immuni alle malattie: nessuno di noi si ammala più o rischia incidenti; quindi, la sera siamo tutti tranquilli che non ci accadrà mai nulla. i pazienti vengono gestiti al Pronto Soccorso da medici e infermieri che fanno il massimo del loro lavoro, ma senza avere gli strumenti idonei. I cittadini non solo soffrono per la malattia o per l'incidente subito, ma soffrono soprattutto un'ingiustizia sociale, che stiamo denunciando ogni giorno in questa

Il Sud è Italia. Immaginate un bambino con una frattura scomposta nell'unico ospedale - oltretutto hanno chiuso il reparto di ortopedia anche a Soverato - che viene stabilizzato con un pezzo di cartone o, una persona anziana con una frattura di femore.

gravissimo che riguarda l'assistenza sanitaria in Calabria ormai da anni: sono undici anni di commissariamento. L'unica nostra speranza è rimasto il viaggio della speranza, ma chi non ha soldi muore. Voi della maggioranza dovete intervenire e porre fine a questo commissariamento: il nostro appello perché vogliamo collaborare per la salute di tutti. Forza Italia chiede questo.

La ragazza, appena ventiduenne, ha riportato una lesione alla cornea, rischiando l'intervento chirurgico. Poche ore prima, sempre nel territorio di Torino, si era svolta una manifestazione di piazza per condannare la recente aggressione ai danni di un altro giovane: uno studente diciannovenne picchiato a sangue in strada perché - cito dalla ricostruzione dei fatti - camminava in modo troppo *gay*. Nemmeno la peggiore dabbenaggine, che è caratteristica alquanto rivalutata ultimamente da certa classe politica, può giustificare chi, come il ministro Salvini, nega l'aumento degli episodi di intolleranza e di discriminazione nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nessuna giustificazione è accettabile di fronte a una deriva tanto ignobile che è invece compito delle istituzioni contrastare con fermezza e rigore. Eppure - quando si dice che non c'è limite al peggio - qualcuno ha provato a giustificare l'ingiustificabile: lo ha fatto il ministro Di Maio - ad esempio - quando in un'intervista ha liquidato l'allarme razzismo in Italia come una montatura della Sinistra contro avviene nel silenzio tombale e assordante del *premier* Conte, l'avvocato degli italiani, ma non di tutti gli italiani evidentemente, non della giovane vittima di razzismo a Moncalieri, non del mio giovane concittadino aggredito perché omosessuale. Eppure, siamo Eppure, siamo innanzitutto noi, care colleghe e colleghi, che abbiamo il compito di agire e di dare il buon esempio: agire sui comportamenti prima ancora che sui reati; agire culturalmente prima ancora che sul piano giudiziario.

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali